*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le politiche europee:* «Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee»

vorrei iniziare il mio intervento con un ringraziamento non formale ai componenti del Gruppo dell'UDC-SVP-Aut (i senatori Cintola - che, tra l'altro, lascia il Senato per tornare all'Assemblea regionale siciliana e che saluto con affetto - Cuffaro, D'Alia, Peterlini, Pinzger, Fosson e Giai) che hanno consentito

senza alcun intento polemico che non era questo il percorso che il Movimento per le Autonomie intendeva avviare per portare alla discussione di questo ramo del Parlamento un argomento tanto delicato: avevo immaginato di coinvolgere in questo impegno gli alleati dichiarati della coalizione di cui il nostro Movimento fa parte.

possibile e, però, rimane integro il valore dell'atto politico e di cortesia istituzionale che il Gruppo dell'UDC-SVP-Aut ha compiuto ritenendo che fosse importante che questo argomento fosse portato all'attenzione del Parlamento. Dopo quella nostra iniziativa tutti gli altri Gruppi parlamentari (il PdL, il PD e l'Italia dei Valori) hanno prodotto atti simili. Devo dire che ‑ probabilmente il dibattito lo renderà chiaro - molte valutazioni sono comuni e attraversano le fila di maggioranza e di opposizione

e le finalità originarie di questo tipo di istituto. Non mi sorprenderò se dovessi verificare in sede di votazione sui documenti delle combinazioni non ortodosse. Già in origine questa vicenda è stata segnata da un certo disordine e, forse, anche da un'incapacità, a cominciare da me, di gestione politica. Non ho mancato di rilevare qualche giorno fa come il Gruppo del PdL, nostro alleato, ha ha rintracciato sul suo documento l'accordo politico molto importante della Lega Nord. Apprezzo questo lavoro perché credo sia costato fatica e intelligenza politica

a relazioni incerte tra i partner di questa coalizione: certo, si trattadi partner di rango diverso, perché la democrazia si fonda sui numeri e comprendo che la esigua rappresentanza del Movimento per le Autonomie determini comportamenti conseguenti. Probabilmente, il giudizio che alla nostra dimensione corrisponda anche la nostra qualità, per cui non c'è da perdere troppo tempo a discutere con il nostro Movimento, neppure delle tematiche per le quali questa alleanza fu sancita: l'alleanza con il nostro Movimento, infatti, fu sancita in quanto venivamo riconosciuti come rappresentanti autentici dell'area territoriale del Mezzogiorno e di un'ispirazione nuova della politica del Governo e delle autonomie in quei territori.

riflessione sintetica che cita soltanto norme relative alla funzione del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), ricorda i riferimenti legislativi che ne vincolano gli impieghi e rammenta al Governo l'utilizzo assolutamente distorto che di tanta parte di quelle risorse

questo Fondo, la cui dotazione in origine è stata intaccata in modo serio per ragioni di finanza pubblica e di compatibilità generale. aveva il compito di stimolare la spesa in conto capitale nelle aree sottoutilizzate - per gran parte nel Mezzogiorno, ma per una parte significativa, anche se residuale, nel Centro Nord

lo sviluppo di quei territori. Era stato coerentemente immaginato un quadro strategico unico tra queste risorse e i fondi comunitari; risorse che si basano sui princìpi della politica di coesione

del Mezzogiorno è stato assolutamente carente. Valga per tutti l'esempio delle grandi agenzie d'investimento, come ANAS e Ferrovie dello Stato, che, attraverso la dotazione che il Tesoro conferisce loro, in questi anni non hanno mai programmato interventi di infrastrutturazione del Mezzogiorno e le uniche risorse che hanno utilizzato

l'elemento di maggiore gravità a cui non si era mai assistito è che nel 2008 e nel 2009 vi è stato un trasferimento secco di risorse destinate al Mezzogiorno a favore di altre aree del Paese, in modo particolare

che non erano oggetto di quel tipo di intervento. Vi è stata poi una grande attenzione alla questione relativa alla quota regionale dei fondi FAS, su cui il Governo ha cominciato ad operare autorizzando la prima *tranche* per la Regione Sicilia; *tranche* solo virtuale dal momento che le prime risorse saranno disponibili nel 2012 e non avendo ancora completato il MISE l'istruttoria per quanto riguarda gli altri PAR regionali: Puglia, Campania e Calabria. di risorse di competenza regionale, mentre quelle su cui si è operato questo meccanismo distorto

sono stati prelevati per incapacità di spesa dei territori del Mezzogiorno è un falso ideologico se non materiale, nel senso che i documenti redatti con queste affermazioni sono falsi. di quanto argomentato chiediamo che il Governo modifichi profondamente il suo indirizzo, ripristini le risorse utilizzate in modo distorto e dia alla politica per il Mezzogiorno un nuovo respiro. Il dibattito ci consentirà di approfondire queste vicende e la dichiarazione di voto finale renderà chiaro qual è il nostro giudizio sulle scelte del Governo.

si è guardato finora come ad una specie di araba fenice della nostra politica economica e finanziaria: talvolta appare e talvolta scompare; talvolta riappare in modo cangiante. come qualcosa di talora troppo pieno e qualche altra volta troppo vuoto; qualche volta, come ricordava l'amico Pistorio, graniticamente indisponibile, qualche altra fin troppo generosamente disponibile ad incursioni (l'amico Pistorio usa il lessico aggiuntivo e sostitutivo che evoca i tempi dell'intervento straordinario). La stessa sensazione rispetto a questo Fondo si ricava ricostruendo in questi anni i nostri lavori parlamentari: i tempi e i modi di approvazione delle nostre leggi, emendamenti e ordini del giorno, proposte del Governo al Parlamento o sollecitazioni al Governo del Parlamento. Per stare in casa nostra, quante volte, all'inseguimento di una parola se non di chiarezza almeno di minore confusione, abbiamo chiesto ad amici e colleghi che tutti stimiamo

il presidente Gasparri e gli altri amici che si onorano di aver sottoscritto questa mozione hanno, in qualche misura, voluto mantenere, a pochi giorni dalla sessione di bilancio - diciamolo chiaramente - nella prospettiva, tra cinque mesi, del rinnovo dei consigli regionali, una mozione

Da quando il lessico dell'amico Pistorio è diventato obsoleto perché non c'era più l'intervento straordinario. Non solo: c'erano i nuovi protagonisti, le Regioni. Fino agli anni Settanta c'era semmai qualche amico di Cuneo Costa nei liberali, Giorgio Bocca su «la Repubblica» - che chiedeva: «ma perché il Mezzogiorno? Ci sono anche le aree depresse del Centro-Nord». Da allora - lo ha ricordato nel suo ultimo intervento in quest'Aula Gerardo Chiaromonte tra tra il 1992 e il 1993 - l'istituto regionale ha tolto alla questione meridionale quel rilievo di grande questione nazionale. Insieme a Gasparri e agli altri colleghi anche della Camera forse qualcuno di voi avrà visto che ieri a Napoli (e lunedì prossimo a Bari)

magari anche a qualcuno seduto sui nostri banchi, è scappata la volgarità: il valtellinese amico di Bossi e Calderoli. No, Tremonti ieri ha detto: il Mezzogiorno non è la somma algebrica delle Regioni meridionali; è qualcosa di più e di diverso. Quindi, un linguaggio valtellinese, come valtellinese era Ezio Vanoni

ha in qualche modo il suo presupposto in quella mattinata di metà luglio in cui alla SVIMEZ abbiamo ascoltato cose drammatiche: la forbice, che nell'epopea di cui ha nostalgia Pistorio si era un po' ristretta, con le Regioni si è drammaticamente divaricata a differenza del ministro Fitto che poté cavarsela con una certa agilità, ebbi la sensazione che la collega Finocchiaro fosse molto appesantita dalla presenza al suo fianco

proprio riferendoci al pessimo uso di queste risorse, richiamato concretamente e crudelmente dai dati del rapporto SVIMEZ, abbiamo pensato - al di là delle formule convenzionali della cabina di regia, dell'Agenzia e così via, non potendo e non volendo, per ragioni di europeismo, restaurare la Cassa per il Mezzogiorno - di dover dare un riferimento politico di coordinamento e di assunzione di responsabilità a Palazzo Chigi; il senatore Pistorio ricorderà infatti che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Io non ho nostalgia della Cassa per il Mezzogiorno, perché la grande stagione della Cassa si è conclusa quando sono arrivate le Regioni. La grande stagione della Cassa risale a quando la Cassa significava geometri, significava ingegneri. Quando ha cominciato a diventare sportello, quando ha cominciato a diventare incentivi non è stata la stessa cosa. Noi vogliamo riportare trasparenza, non solo sui fondi, ma anche sul nostro modo di lavorare, su quel fondamentale istituto di democrazia che è il Governo in Parlamento. abbiamo anche sfidato l'ironia. L'abbiamo fatto volutamente, impegnando il Governo a predisporre un piano per il Mezzogiorno. Collega Finocchiaro, perché abbiamo sfidato l'ironia? solito il piano non fa parte, come lessico, del bagaglio di centrodestra, fin troppo appesantito da liberismi di maniera. Perché il piano, nel senso del documento elaborato

Priorità è compatibilità, perché altrimenti il "mezzogiornismo" diventa vittimismo, diventa gargarismo fine a se stesso, e allora ci vuole quella responsabilità politica che ci ha portato ad indicare soluzioni. Collega Pistorio, ci conosciamo abbastanza: nel mio stato d'animo, tra i piccoli e i grandi sono sempre stato con i piccoli. Voi avevate presentato un testo pienamente compatibile con il nostro, sotto i colpi del vento del partito del Sud. Il nostro punto di vista, invece, non voleva assolutamente essere confuso allora con questo vento. Ma non abbiamo alcuna preclusione. Probabilmente si potrà rilevare come le impegnative siano abbastanza simili. Credo, signor Presidente, di aver assolto il mio compito,

un economista vero e serio, che ha detto, sul fiume di risorse del perverso e distorto regionalismo all'italiana, quel che si doveva dire dai banchi del centrosinistra. *(Applausi dal Gruppo PdL.

dal momento che li ha disattesi tutti, anche quelli solennemente annunciati e confermati nel corso dei dibattiti e degli incontri con le forze economiche e sociali, quanto ad affrontare il tema dell'Italia. Quello che abbiamo di fronte non è solo il problema della sottrazione di risorse al Fondo aree sottoutilizzate. infatti con tutta evidenza l'assoluta mancanza di una politica per il Paese, di un'idea circa la funzione che questo Paese deve esercitare in Europa e nel mondo, circa la circostanza che vede l'Unione europea, che conta qualcosa, a parere di taluni, orientare le proprie politiche e le proprie scelte in direzione dell'area di futuro libero scambio, che riunisce centinaia di milioni di cittadini che condividono con noi un'area importante, il Mediterraneo. una politica in relazione alla capacità di cogliere le opportunità che abbiamo di fronte. Ci vengono dispensate banalità.

di apertura, di liberalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, non già per realizzare mercati contendibili (che sarebbe audace sperare da parte di questa maggioranza), tentare di realizzare il minimo indispensabile di modernizzazione del nostro Paese e della pubblica amministrazione. Oggi si vuole dire che la grande rivoluzione è annullare la pubblica amministrazione, destrutturare le istituzioni e non già occuparsi del problema del loro funzionamento. Si dice questo mentre si assume che sia necessario in questo momento enfatizzare le capacità regolatorie dei Governi e della politica.

che puntano semplicemente a «passare la nottata» nel mentre si saccheggiano le risorse pubbliche (non le risorse del Mezzogiorno, ma quelle pubbliche) per ripianare i bilanci di Comuni male amministrati, dando prova che la cattiva politica e la cattiva amministrazione vengono premiate per spostare risorse su settori improduttivi e assistenziati. abbiamo il timore che il federalismo fiscale possa rispondere a due esigenze, entrambe di natura politica: da una parte, assecondare le pulsioni dell'egoismo sociale e territoriale e, dall'altra, soddisfare attraverso altre modalità la domanda di assistenza e di trasferimento di risorse pubbliche prive di regole, di finalizzazione e di capacità di verifica e di controllo, e di controllo, funzione che compete alla pubblica amministrazione e alle consapevoli politiche pubbliche che devono regolarla. Il problema che abbiamo di fronte è esattamente questo, non ci si venga a dire che i soldi fanno male. Sappiamo che i soldi quando sono male utilizzati fanno male, ma qualcuno ci venga a spiegare com'è possibile garantire legalità e sicurezza nel Mezzogiorno se non attraverso investimenti in conto capitale e in conto gestione. Qualcuno ci venga a spiegare com'è possibile fare del Mezzogiorno un luogo di attrazione per la formazione delle nuove classi dirigenti nell'area euromediterranea, senza conseguentemente investire nei centri di ricerca pubblici e privati, da finanziare in base a criteri obiettivi di merito e di verifica dei risultati. Qualcuno ci venga a spiegare com'è possibile realizzare condizioni di civiltà per garantire il minimo di operatività ai cittadini e alle imprese, ad esempio nel sistema della logistica e dei trasporti, senza investire le risorse finanziarie necessarie per realizzare questi obiettivi. Allora il problema non è spendere bene o male le risorse pubbliche, perché le risorse pubbliche vanno spese sempre bene ed è dovere dello Stato potenziare e rendere efficienti e efficaci i sistemi di controllo, nonché affinare i meccanismi procedurali affinché fisiologicamente possano essere evidenziati i fattori distorsivi che dovessero emergere nell'applicazione degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Noi tentiamo di richiamare l'attenzione del Governo su questi problemi perché la situazione del Paese e del Mezzogiorno ormai è al limite.

che imponeva la costituzione di una rigida cabina di regia affinché gli investimenti a titolarità regionale fossero

Quella cabina di regia non è stata costituita, nonostante la legge n. 296 la prevedesse espressamente, così come si disattende sistematicamente l'addizionalità della spesa nel Mezzogiorno e si destruttura il Quadro strategico nazionale 2007-2013. Ma tanto che cosa ci importa dell'Europa e della decisione comunitaria! Si può sempre dire

Noi ci batteremo per il Mezzogiorno e per questo chiediamo al Governo di rispettare gli impegni indicati nel nostro documento, perché questo fa bene all'Italia e al Mezzogiorno e garantisce i diritti di cittadinanza in tutto il Paese.

Le ragioni per le quali l'Italia dei Valori ha presentato questa mozione le abbiamo già spiegate nel corso dei lavori delle Commissioni parlamentari, soprattutto in occasione della valutazione del decreto-legge n.

Per noi e per il Paese è una questione centrale, se pensiamo che le risorse del FAS, stanziate con la finanziaria per il 2003 e modificate poi con quella per il 2007, sono lo strumento prevalente di finanziamento, insieme a risorse aggiuntive nazionali, delle politiche di sviluppo per le aree sottoutilizzate del Paese (una definizione, questa, che è un timido eufemismo con il quale si indicano in sostanza le Regioni povere e le aree in crisi industriale). I principi che avrebbero dovuto regolamentare l'utilizzo di queste risorse, dunque, erano quelli del finanziamento degli obiettivi di riequilibrio economico e sociale e della addizionalità delle risorse, che non possono sostituirsi a quelle della politica ordinaria. La sostanza del problema di cui stiamo discutendo oggi è che i circa 65 miliardi che rappresentavano la dotazione iniziale dovevano essere destinati a progetti regionali o parzialmente statali aggiuntivi rispetto alla spesa ordinaria e finalizzati ad interventi che avessero lo scopo di diminuire il dislivello tra territori ricchi e poveri. Ebbene, di quei 65 miliardi iniziali, circa 13 miliardi sono stati utilizzati, fino al 2008, per la copertura di leggi, per cui le risorse destinate alle Regioni sono ormai ridotte, forse,

Si trattava di soldi destinati da anni allo sviluppo meridionale, ma utilizzati come cassa per qualsiasi intervento, da quello della banda larga al risarcimento a favore degli obbligazionisti Alitalia. sono in un certo senso debiti statali verso le Regioni e non interventi aggiuntivi, come si è cercato di far credere in alcune comunicazioni. si comprende il malcontento sempre più diffuso tra le istituzioni meridionali dato che il Governo promette per domani finanziamenti che si sarebbe dovuto iniziare ad erogare già da due anni. Numerose sono le partite aperte che hanno determinato dal 2 luglio l'interruzione dei rapporti istituzionali tra Governo e Regioni, per la prima volta nel nostro Paese, e i nodi del contendere restano sempre in sospeso. Non solo le risorse del FAS, ma anche il Patto per la salute 2010-2012, con i 7 miliardi di fabbisogno aggiuntivo stimati, e poi la scuola ed il turismo. Il Governo, e noi non avevamo dubbi al riguardo, dimostra di essere poco credibile. Dopo che il FAS nazionale è stato usato per coprire spese correnti e dare contributi ai Comuni di amministrazioni amiche, come Roma, Catania e Palermo, ora si chiede di rimodulare anche la quota regionale dopo l'accordo di febbraio e dopo la delibera CIPE del 6 marzo, cosicché se il Governo può partire dal non speso sta ancora una volta sbagliando di grosso, in quanto le risorse in buona parte sono state già programmate e in diversi casi impegnate dalle Regioni: se immagina una centralizzazione della programmazione, non solo compie un errore di prospettiva ma va in una direzione opposta al federalismo. In sostanza, nessuna risorsa aggiuntiva è stata messa a disposizione da questo Governo - deve essere chiaro - e si sta ancora facendo riferimento esclusivo a risorse stanziate dal centrosinistra di Prodi. Allo stesso modo nessun serio programma di sviluppo collegato alla scadenza della legislatura è stato elaborato e sostenuto da questo Esecutivo. Anche questo deve essere chiaro. Insomma, niente di niente. Il Ministro dell'economia di certo obietterà che con una crisi economica di queste dimensioni nessun Governo sarebbe stato in grado di reperire risorse, ma resta la palese contraddizione, il punto dolente, che di fronte alla necessità di una maggiore attenzione al Mezzogiorno, la gran parte dei provvedimenti anticrisi è stata finanziata con fondi che per legge, per una quota pari all'85 per cento, spettavano alle Regioni meridionali, ossia quelle più esposte agli effetti devastanti della crisi. Qual è il risultato prodotto? In primo luogo, sono diminuite le risorse per investimenti infrastrutturali, nonostante il Governo già con la manovra d'estate avesse manifestato l'intenzione di destinare le risorse FAS riprogrammate in via prioritaria ad interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Paese. A quasi un anno di distanza, la metà delle risorse finora riprogrammate sono state utilizzate per finanziare spese correnti e di gestione, come i contratti di servizio di Trenitalia, la privatizzazione della società Tirrenia SpA, l'adeguamento prezzi, di modo che i finanziamenti assegnati sono inferiori a quelli inizialmente previsti. luogo, le risorse FAS non sono state riprogrammate in chiave anticiclica destinando, come avevamo noi richiesto, una quota rilevante delle risorse ad un piano di opere medio-piccole diffuse sul territorio e quindi immediatamente cantierabili e capaci di dare un segnale di operatività

nei prossimi mesi sono incerte, tant'è che è comprensibile l'opposizione delle Regioni al ridimensionamento delle quote relative ai programmi FAS ed è legittimo il loro sospetto. La questione meridionale, di cui tanto si è parlato, da questione nazionale sta sempre più diventando - con i decreti che il Governo sta formulando - un carrozzone mediatico, un tormentone aggrovigliato, e sta mettendo in moto azioni e reazioni i cui risultati finali sono ancora oggi del tutto imprevedibili. La questione meridionale - lo ripetiamo per l'ennesima volta - non è solamente questione di risorse economiche, ma soprattutto di strategia di politica economica o, meglio, giudicando quello che sta facendo il Governo, della completa assenza di una politica economica per il Sud. Nessuno qui vuole difendere il partito della spesa del Sud, che usa le risorse per creare e mantenere clientele elettorali, ma vogliamo solo prendere atto allo stato attuale di una assoluta mancanza di politiche per il Mezzogiorno, perpetuata consapevolmente e coscientemente da questo Governo. Se a livello territoriale esiste un problema di qualità degli amministratori che governano le Regioni meridionali, la soluzione non è però il raschiamento di risorse, ma quella di vigilare sull'utilizzo di queste sul piano politico, facendo pesare responsabilità individuali, come stiamo facendo noi per quanto riguarda le nostre responsabilità di giudizio, anche, laddove è necessario, sul piano giudiziario. Il Governo non appare legittimato a criticare la polverizzazione degli investimenti e il ritardo nella esecuzione delle opere pubbliche, quando la legge-obiettivo nazionale si sta dimostrando incapace di calendarizzare e rispettare i tempi. E soprattutto, dopo che, per la prima volta da dieci anni a questa parte, nei DPEF varati dal Governo Berlusconi non si fa alcuna menzione della ripartizione territoriale della spesa totale in conto capitale per il Mezzogiorno, questo Governo si dimostra incapace di offrire al Paese una visione complessiva e unitaria di quanto ha intenzione di fare. Ragionando in termini di cassa, per accontentare il Governatore della Sicilia, occorrono circa 4 miliardi altri 3 per assicurare la copertura del Programma attuativo regionale della Puglia. In Abruzzo il ministro Matteoli, pochi mesi fa, ha annunciato l'Atto aggiuntivo dell'Intesa generale quadro con infrastrutture per oltre 3 miliardi, di cui 1,7 di investimenti nel prossimo triennio. E nella stessa situazione sono tutti i Programmi attuativi regionali delle Regioni meridionali, mentre hanno già ottenuto la prima approvazione del CIPE la gran parte delle Regioni centro-settentrionali. I fondi FAS hanno subito una evoluzione della specie. Lo dico con serenità e senza polemica: da pozzo di San Patrizio si sono prima trasformati in un gioco abile delle tre carte e poi, a beneficio degli ingenui e per la tranquilla sopravvivenza della maggioranza, in un'opera di illusionismo. Nasceva così alcuni mesi or sono il cosiddetto piano Berlusconi. L'obiettivo era di individuare con una cabina di regia i progetti cui destinare i fondi FAS. Erano stati assicurati soldi alle Regioni, con una gestione da parte della Presidenza del Consiglio attraverso una cabina di regia composta dai Dicasteri che concorrevano al piano. A complicare le cose, è sopraggiunto il braccio di ferro in corso nella maggioranza e nel Governo. Restano - per rifare un po' di conticini - meno di 5 miliardi che dovrebbero accontentare le esigenze dei Ministri finora esclusi o penalizzati dalla lotteria della redistribuzione: in prima fila, lo stesso Scajola e poi il Ministro dell'istruzione, e poi ancora quello dell'ambiente, quello delle politiche agricole. Ora apprendiamo, per la soddisfazione dei partecipanti a un convegno, che è nato il piano Tremonti che presenta lo studio di tre idee per rilanciare il Sud: una rivoluzionaria, volta ad utilizzare i depositi fiscalmente agevolati per gli impieghi nel Meridione, dopo che si era rinunciato alla fiscalità di vantaggio con la eliminazione della Visco-Sud; una fantasiosa, con il potenziamento del CNR con i fondi europei, dopo i tagli lineari consistenti alla ricerca e alla innovazione; infine, una riciclata, come la Banca del Sud, con la speranza che almeno questa, nella politica creditizia, abbia più fortuna dei Tremonti *bond*. Per queste ragioni, con un sussulto di speranza per il nostro Paese, noi dell'IdV chiediamo, chiediamo, con questa mozione, impegni precisi del Governo, augurandoci che questo sussulto di speranza non si trasformi in uno stillicidio per il Sud.

aspettati da parte delle forze facenti parte di questa maggioranza, era un atteggiamento di soddisfazione, di esultanza e anche di raggiungimento di alcuni obiettivi prefissati con

i fondi destinati alla Sicilia stessa attraverso i fondi FAS. Invece, ancora una volta, anticipato certamente anche da chi ha potuto seguire le agenzie o gli articoli di stampa, si assiste ad una mistificazione e a una strumentalizzazione della battaglia sui fondi FAS. Tutto questo, ormai, è abbastanza chiaro e anticipa una posizione politica nota.

allo scoperto: non tanto per coerenza e dignità nei rapporti politici con gli altri alleati ma, soprattutto, per rispetto del voto chiesto ai siciliani e alle

salvo il fatto di avere assunto delle posizioni chiare e intransigenti rispetto al ruolo dello Stato nei confronti delle Regioni del Sud che certo - e di questo chiedo scusa, da siciliana, all'Italia intera - non hanno dato uno spettacolo

chiarezza e smettere di stare con due piedi in una scarpa. Non si fa così politica, perché la vostra è caratterizzata da doppiogiochismo, da ambiguità e da inaffidabilità. Il doppiogiochismo lo vediamo certamente nel fatto che, rispetto ad un programma e a degli obiettivi che, come dicevo, si sono dati al proprio popolo, si offende la volontà degli elettori che li hanno votati. L'ambiguità è perché siete al Governo nazionale, nonostante un articolo dell'MPA, pubblicato il 27 settembre, minacci ancora una volta,

e non all'alleanza con la quale l'MPA si è presentato al cospetto degli elettori. Inaffidabili perché vi smentite da soli. Voglio qui ricordare come, appena il 24 settembre venisse ringraziato e molto apprezzato il ministro Scajola per lo sblocco dei fondi FAS e come poi, il 27 settembre, venisse minacciata ancora una volta la fuoriuscita dal Governo.

di sentirsi dire che le risorse destinate al Sud vengono sprecate perché mancherebbero le energie positive e la capacità di utilizzarle al meglio,

Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, nell'affrontare la questione del Mezzogiorno vorrei partire da un riferimento all'attualità: l'approvazione qualche giorno fa, in quest'Aula, dell'emendamento, al decreto-legge anticrisi, che estende la copertura dello scudo fiscale anche per i capitali i cui titolari sono accusati di falso in bilancio. Un atto grave che, come ho avuto modo di dichiarare, segna la legalizzazione dell'illegalità. Altro che pacchetto sicurezza! Al di là dei proclami di Berlusconi e dei suoi Ministri sulla lotta alla mafia e al riciclaggio, questo emendamento mette a rischio la sicurezza e la tenuta democratica del nostro Paese. Nel Governo è prevalsa ancora una volta la logica dei condoni, avvantaggiando chi ha evaso la legge a scapito di quanti negli anni hanno pagato le tasse. Così si alimentano le disuguaglianze in un Paese già fortemente sperequato. A farne le spese, infatti, saranno i cittadini onesti che, a costo di sacrifici, hanno sempre fatto il loro dovere e, al solito, le aree più deboli. Se realmente si vuole affrontare la questione Mezzogiorno, che poi è una questione nazionale, bisogna pensare a combattere la criminalità organizzata, in tutte le manifestazioni che essa si dà: ed è una battaglia, questa, che deve sostenere la politica. È la politica che deve definire la cornice nella quale, attraverso le istituzioni e il coinvolgimento delle forze sociali, collocare gli interventi di programmazione economica, le iniziative imprenditoriali, gli investimenti per scommettere su un futuro di legalità prima di tutto per i nostri giovani. Il lavoro di controllo, repressione e indagine che quotidianamente svolgono le forze dell'ordine e la magistratura è fondamentale, ma rischia di rivelarsi insufficiente senza il necessario apporto e la doverosa attenzione della politica, alla quale spetta il compito di creare le condizioni per cambiare la marcia e offrire, soprattutto alle giovani generazioni, la speranza di un destino diverso. Ebbene, di fronte a questo stato di cose, che lacera il tessuto sociale della comunità, alimentando timori e incertezze negli ambienti imprenditoriali, allontanando le opportunità di sviluppo, qual è la risposta del Governo? Tagliare le risorse del Fondo destinato alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno. Questa è la prova che il centrodestra ritiene il destino del Sud immodificabile, il dilagare della criminalità inevitabile. E invece no, onorevoli colleghi, dobbiamo dire forte e chiaro che non può essere così. Per questo chiedo che il Governo ripristini i circa 30 miliardi di risorse dei fondi FAS, fino ad oggi sottratti al Mezzogiorno. Quei fondi servono per creare opportunità di sviluppo: i fondi FAS possono rappresentare una straordinaria occasione per gettare le basi di uno sviluppo strutturale mediante il potenziamento dei servizi. sull'offerta dei servizi che oggi si misura la competitività di un territorio? In tema di servizi, come tralasciare il riferimento all'emergenza rifiuti, che ha messo in ginocchio la Campania, ma rischia di esplodere anche in altre Regioni meridionali? della Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le attività illecite ad esso connesse, anche sulla base delle dichiarazioni rese da amministratori, imprenditori del settore e magistrati relative alla fortissima invadenza delle organizzazioni criminali nel settore dei rifiuti è emblematico, da ultimo, il caso delle navi dei veleni affondate al largo delle coste tirreniche - sono sempre più convinto che una delle vie di uscita da una situazione che vede la politica e le istituzioni in forte ritardo rispetto all'avanzata delle mafie sia la redazione di una legge quadro sul ciclo integrato dei rifiuti, cui siamo chiamati anche a livello europeo con il «Pacchetto 20-20-20». Stabilire, con una legge specifica, regole chiare per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti vuol dire scrivere la parola fine sotto il capitolo dei commissariamenti, facendo prevalere, su quella della delega in bianco dettata dall'emergenza, la logica della programmazione condivisa, della responsabilità e della responsabilizzazione della classe dirigente; vuol dire fermare con la forza della legge il dilagare della criminalità, garantendo in tal modo la sicurezza collettiva e

e non un commissario straordinario di tanti frammenti che rispondono a interessi particolari. Bisogna invertire la rotta per trovare soluzioni concrete, per far uscire il Mezzogiorno dalla crisi che lo attanaglia con una profonda conversione culturale.

oggi, prendendo spunto da ciò che ha detto poc'anzi il collega De Luca, materiale e geografica collocazione: essa giace sui fondali di Cetraro ed è meticolosamente suddivisa in fusti di scorie nocive; giace nei campi di Castrovillari e della Sibaritide; giace ancora sul territorio di Crotone dove ha operato l'ex Pertusola. Questi episodi mi offrono l'occasione, signor Presidente ed onorevoli colleghi, per un rapido esame dello stato della legalità nel nostro Paese, di quella cultura della legalità che permea tutta la mozione presentata dal Partito Democratico. Il nostro Mezzogiorno non è neppure privo di strumenti per il sostegno allo sviluppo, tra i quali l'ingente flusso di fondi strutturali comunitari, i fondi FAS, la legge n. lo sforzo, per quanto ponderoso, rischia di perdersi in mille rivoli, asserviti al particolarismo ed ai bisogni localistici. È evidente che anche l'azione pubblica, l'impegno delle energie positive del Mezzogiorno non impediscono la devastazione dell'ambiente, il saccheggio delle risorse, l'appropriazione esclusiva ed escludente di beni universali. Non impediscono il prodursi di un danno oltraggioso di dimensioni difficili da prevedere al momento. un danno prodotto dal desiderio ingiusto di pochi di arricchirsi alle spalle e sulle spalle dei molti che cercano una convivenza pacifica ed ordinata. DE SENA). Perché? Cosa manca per raggiungere un punto di corretto equilibrio tra il legittimo interesse individuale ed il benessere collettivo? Qual è il tassello che serve a completare un quadro di relazioni rispettose dei principi universali prima che delle leggi e dei regolamenti? È qui che gli strumenti di intervento non dotati di una coscienza rispettosa dell'agire etico mostrano i loro limiti. L'idea che il contemperamento degli interessi particolari possa derivare in prevalenza dall'incremento incondizionato dei mezzi di produzione, e quindi di arricchimento, pare mostrare i suoi limiti, come la recente crisi finanziaria globale ci insegna. L'accentuazione delle capacità prestazionali a discapito di una visione valoriale che ponga l'uomo al centro del mondo genera tensioni competitive malsane in virtù delle quali qualunque fine, purché di arricchimento, giustifica qualunque mezzo per raggiungerlo. Così nascono le scorie dell'era moderna: scorie etiche prima che industriali. Ancora una volta lo si vede dal dibattito generale: è il Sud sul banco degli imputati. Ancora una volta si confonde il cinismo predatorio delle organizzazioni criminali con la rassegnazione di genti fiaccate da decenni di malaffare, inefficienza della pubblica amministrazione, assenza di risposte concrete da parte della classe politica. Tutta la classe politica. Ancora una volta si afferma il principio che al Sud c'è un problema del Sud e non dell'intero Paese. Questo è sbagliato. È sbagliato in genere poiché l'unitarietà geografica e politica implica un impegno a tutto campo di qualunque forma di Stato, sia esso federalista o meno. Ma è soprattutto sbagliato nella specie, poiché la colpa dell'ennesimo stupro della terra meridionale ricade anche sulle spalle di chi, grazie all'intervento illecito di banditi senza scrupoli, lo ha originato. Infatti, da dove vengono queste scorie? Chi ha alimentato questo oscuro e - a quanto pare - molto esteso traffico di nocività? Chi può invocare ad esimente la mancata conoscenza delle qualità e della quantità dei veleni riversati nel mare di Calabria e chissà dove altro? domande pesanti, alle quali si spera che gli inquirenti diano un risposta. Ma se anche essa arriverà, non sarà certo compito degli inquirenti ricostruire la trama e l'ordito di una relazione corretta tra il Nord e il Sud del Paese. Nell'individuare il contesto nel quale ha potuto crearsi il problema, non intendo accentuare le divaricazioni esistenti tra Nord e Sud per mezzo di una naturale quanto scontata chiamata in correità del mondo produttivo. Si sa, chi produce, trasforma e distribuisce tende ad ottimizzare i propri cicli di lavorazione e di scarto e mira alla realizzazione del massimo profitto con il minimo sforzo. È l'economia moderna. Tuttavia, un Paese che - secondo stime prudenti - accetti che una consistente quota annua di milioni di tonnellate di scorie più o meno nocive, derivanti da processi di lavorazione industriale, sia smaltita con patti scellerati deve fare molta strada in termini di solidità dell'impianto etico, giuridico e amministrativo. Esistono, con evidenza, vuoti di tipo amministrativo; mancano le sensibilità nella politica e nell'amministrazione (evidentemente, fatta eccezione per alcuni, nobili casi). Si corre ai ripari solo in presenza del danno, una volta scoperto, ma il vuoto vero da colmare è, *in primis*, nell'agire morale. Presidente, mi avvio alla conclusione, ritenendo che oggi il tema dello sviluppo del Mezzogiorno si leghi indissolubilmente ad alcuni nodi chiave per il futuro del nostro Paese sulla scena globale, primo tra essi il dissolvimento dei neoparticolarismi e del dualismo Nord‑Sud in un unico movimento virtuoso nazionale. In secondo luogo, è necessario impedire che la dicotomia tra un Nord produttivo ed un Sud sicuramente capace di recuperare il proprio ritardo, ma intriso della subcultura dell'illegalità possa fornire alibi di comodo a tutti coloro che desiderano che tutto cambi perché nulla cambi, ad iniziare dalla classe politica ed amministrativa di questo Paese. una vera e propria inversione dei poli della dialettica politica, cercando di tornare all'alto di una politica di programmazione, piuttosto che permanere al basso di una politica di minutaglie. In terzo luogo, bisogna rompere l'assedio ideologico delle menti dei cittadini che vedono comunque nello *status quo* una modalità accettabile, pur se non gradevole, per realizzare la convivenza nei territori di residenza. In quarto luogo, partendo dal rispetto dell'altro, occorre consolidare nei giovani la coscienza del rispetto dell'ambiente naturale e della vivibilità del contesto globale come teatro del confronto, del dialogo e del dibattito politico, sociale e culturale nel prioritario interesse collettivo. Infine, signor Presidente ed onorevoli colleghi, ritengo che i recenti accadimenti calabresi siano un oltraggio all'ambiente non solo naturale, ma soprattutto globale del sistema Paese, e non soltanto meridionale, nel quale insiste un'inquietante fascia grigia di connivenze e di contiguità con il movimento mafioso affaristico, sul quale la politica, l'alta politica di questo Parlamento deve intervenire con estrema decisione e altrettanta lungimiranza per snellirne sistemicamente la portata fino ad annullarla.

il senatore De Sena ha giustamente ricordato che continuiamo a parlare di una questione meridionale che dura da troppo tempo nel Paese.

Sarebbe veramente triste immaginare di continuare a parlare di questa nuova questione meridionale - se vogliamo chiamarla così, perché la guardo in rapporto al Paese che vogliamo, che è l'Europa - ancora per i prossimi sarebbe certamente triste per il Meridione e per il Mezzogiorno, per averla subita per tanto tempo in questi anni, ma rischierebbe di diventare triste per tutti, soprattutto per l'Italia, portarsi ancora dietro una vicenda di questo tipo. Tuttavia, ho l'impressione che le politiche economiche di questi ultimi mesi siano tutte orientate a far rimanere il Mezzogiorno del nostro Paese ancora

stiamo ridistribuendo a nostro uso e consumo i fondi FAS, che dovrebbero essere destinati allo sviluppo infrastrutturale del Mezziogiorno, ma perché dietro la la scelta del Governo nazionale di distribuire tali fondi c'è la negazione della politica federalista, cari amici della Lega. Non si può volere con forza e con determinazione, così come avete desiderato voi, una legge sul federalismo e poi consentire al Governo del quale siete parte importante di distribuire le risorse che per legge, invece, vanno assegnate alle Regioni assegnate alle Regioni che dovrebbero programmarle. È un controsenso: è la prima norma federalista che dovremmo avere il coraggio di rispettare, quella che da qualche anno sta funzionando. Sono stato per tanti anni Presidente di Regione e non mi era mai capitato che il Governo nazionale programmasse i fondi FAS, che sono fondi delle Regioni! *(Applausi del che li stiamo stornando o no, che è già grave di per sé: la cosa più grave per un Governo che ha voluto una legge sul federalismo è programmare risorse che invece andrebbero date alle Regioni e che le stesse Regioni dovrebbero programmare.

giusta, che noi condividiamo e che vogliamo, ma vorrei soltanto ricordare al senatore Pistorio che in questo anno e mezzo non è stata spesa una sola lira

che i bandi fossero pubblicati oggi, si potrebbe cominciare ad attivare la spesa tra un anno. Ma la Sicilia al 31 dicembre disimpegna oltre un miliardo di euro, questa è già una certezza perché non ci sono i bandi, per cui non si può neanche discutere se dovranno essere o no giustificati come spesa. Allora, capisco quanto sia complicato affidare ad una Regione come la Sicilia la possibilità di portare avanti una norma sul federalismo, che non abbiamo condiviso ma che, essendo una legge di questo Parlamento, abbiamo il dovere di rispettare, quando il Presidente della Regione, piuttosto che farsi garante dello sviluppo e della responsabilità di una legge che è stata voluta, continua ad utilizzare tutto ciò di cui dispone mettendolo al di sopra delle istituzioni e facendo piuttosto gli interessi del suo partito. Capisco che è difficile dover tentare di rappresentare questo purtroppo in questi anni sono tutte contro il Mezzogiorno. Per citarne soltanto una: vi siete resi conto di cosa significano le politiche agrarie per questo Paese nell'ultimo anno e mezzo? Senatore D'Alia, lei lo sa che cosa sta succedendo in Sicilia nel reparto vitivinicolo?

ed il motivo è molto semplice: le cantine non comprano l'uva perché hanno i serbatoi pieni. E i serbatoi sono pieni perché questo Governo, insieme all'Unione europea, ha cambiato la politica agraria

il gioco è servito: quest'anno in Sicilia il sistema vitivinicolo sarà al collasso. Aggiungeteci il problema del grano e dell'olivicoltura; in cambio, dall'altra parte, abbiamo varato una bella legge legge sulle quote latte. Credo che non soltanto i fondi FAS, ma bisognerebbe avere il coraggio di rivedere l'intera politica sul Mezzogiorno perché sta penalizzando la Sicilia e non aiuta certo l'assunzione di responsabilità.

ieri a Napoli abbiamo assistito ad una *performance* di alcuni rappresentanti del Governo e di alcuni colleghi della maggioranza che hanno organizzato e partecipato ad un convegno sulla questione meridionale. Se posso permettermi una battuta, Napoli è abituata alle sceneggiate, ne sa apprezzare anche il lato artistico. Quella di ieri è una *performance* che definire inutile è un eufemismo. Preceduto da un'intervista concessa a «Il Mattino», il ministro Tremonti ci ha raccontato la sua ricetta per «salvare il Mezzogiorno» perché - cito le sue parole - «proprio il rilancio del Meridione è una delle priorità del Governo per far ripartire l'economia». il Ministro ha snocciolato la sua ricetta: le zone a burocrazia zero, il Consiglio nazionale per la ricerca, la Banca del Sud. E il ministro Brunetta ci ha rassicurati che il piano per il Sud sarà «tutto verticalizzato su Berlusconi e Palazzo Chigi e Palazzo Chigi per vincere la grande sfida per il Mezzogiorno già nei prossimi mesi e non nell'arco di 5-10 anni». A parte qualche considerazione nel merito delle proposte (sono state approfondite molto bene dal collega Bubbico), alcune delle quali sono un po' estemporanee, viene da chiedersi se siamo stati e siamo nello stesso Paese e nello stesso Parlamento, se quelle parole e quelle proposte arrivano da Ministri dello stesso Governo che ha mortificato e penalizzato le terre del Mezzogiorno in questo primo anno e mezzo di legislatura. Viene da chiederci - e non pensate che i cittadini napoletani o i campani o i meridionali non se lo chiedano - chi vi ha impedito di fare le cose che dite di voler fare. Se qualcuno ve l'ha impedito

Maggioranza e Governo fino ad oggi hanno solo tagliato fondi (è stato ripetuto tante volte: lo scippo dei fondi FAS) per miliardi e miliardi di euro. Soldi finalizzati allo sviluppo delle aree sottosviluppate che sono stati stornati colpevolmente iniziative meritevoli, come ad esempio l'Abruzzo. Avremmo dovuto dirlo, però, ai cittadini meridionali che essi da soli dovevano compiere questo sforzo di solidarietà nei confronti di quella terra martoriata. stati utilizzati anche per l'ICI, per permettere alle persone che possono permetterselo (per esempio, un parlamentare) di non pagare più questa Abbiamo cercato noi di difendere il Sud in quest'Aula, di ripristinare strumenti per lo sviluppo, per il lavoro, per facilitare la vita delle imprese. Lo abbiamo fatto in ogni provvedimento, cercando anche di di attirare l'attenzione con interrogazioni ed interventi in Aula su questioni drammatiche del nostro territorio. Penso alla mia Regione, al caso Pomigliano, alla Fincantieri: questioni drammatiche che il Governo ha voluto derubricare a tavoli tavoli tecnici, a questioni affrontate solo da dirigenti. Solo no e solo tagli. Parlare oggi, come fa il ministro Tremonti, di fiscalità di vantaggio, dopo aver smantellato gli strumenti di fiscalità di sviluppo, suona, come ha detto la Capogruppo, senatrice Finocchiaro, come una presa in giro. Solo un *bluff*. Solo fumo. Solo chiacchiere. La maggioranza ed il Governo sul Sud non hanno né volontà di azione né veri programmi e sbandano tra tagli, penalizzazioni e suggestioni di irrealizzabili partiti del Sud da contrapporre ai forti partiti del Nord. Siamo fermamente convinti che quella meridionale, così come ci hanno insegnato Giustino Fortunato e Manlio Rossi Doria, sia una grande questione nazionale e che in questo modo vada affrontata. Si tratta di un grande confronto che necessariamente dobbiamo aprire tra di noi, qui, in Parlamento. È la politica che deve riappropriarsi della questione meridionale. Se si vuole riparlare seriamente di Sud si riparta da una seria analisi delle condizioni in cui vive oggi quell'area. Il recente rapporto SVIMEZ - lo abbiamo già ricordato in quest'Aula - è molto chiaro in questo senso. Vi si segnala la grave situazione della Campania, dove nel 2008 si è registrata una diminuzione del PIL particolarmente elevata (2,8 dove nell'ultimo anno hanno chiuso le saracinesche più di 1.000 negozi di abbigliamento, dove un laureato su due emigra, va via. Dobbiamo ripartire anche dal richiamo autorevole che hanno fatto oggi i vescovi, come fecero vent'anni fa con un documento che andrebbe riletto anche oggi. Smetterla con il silenzio sul Mezzogiorno! La nostra mozione va in quella direzione. Propone un nuovo progetto nazionale sul Mezzogiorno, per la sua crescita, per la valorizzazione delle sue potenzialità. Un progetto che si rivolga alle piccole e medie imprese che si espongono ai rischi dell'internazionalizzazione, che hanno imparato i vantaggi della rete, specialmente nell'utilizzo dell'innovazione e delle nuove tecnologie. Un progetto che sostenga tecnologie. Un progetto che sostenga il Sud eccellente. I nostri centri di ricerca, pubblici e privati, raggiungono livelli altissimi, malgrado lo scarso aiuto da parte dello Stato. Vi sono imprese che hanno imparato a dialogare con le università e che investono nella spesa in ricerca e sviluppo, dall'indagine di UniCredit. Dunque, non un apparato produttivo solo in attesa di finanziamenti pubblici. però è un processo incompleto, che rischia di interrompersi bruscamente e di bruciare esperienze molto positive, che invece hanno bisogno di concreti piani di investimenti pluriennali, per esempio per ridurre il *digital divide*. In proposito, il Governo Prodi aveva iniziato un cammino molto interessante, poi tutto si è bloccato. Un Sud moderno che vuole, accanto alla necessità di superare atavici problemi, anche sperimentare percorsi di modernità.

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ho ascoltato e partecipato a questo confronto maggioranza. È un argomento importantissimo, perché è vero quello che dice il ministro Tremonti:

non è questione di oggi, della crisi o dell'anti-crisi: la questione meridionale c'è da prima della Cassa per il Mezzogiorno. È una questione che i meridionali non sanno risolvere. Voi chiedete sempre l'aiuto del Governo, bisognerà forse rimboccarsi le maniche e darsi veramente da fare, con l'aiuto del Governo. Anche la categoria sociale del Meridione si deve dare da fare. Vengo dal Consiglio regionale dell'Umbria, regione governata dalla sinistra.

in cui si vive abbastanza bene e in cui si lavora. Quando usufruivamo dei fondi comunitari, verso il quinto anno, prima della nuova programmazione,

significa non avere idea di che cosa fare con le risorse e le provvidenze che lo Stato ti mette in mano. Mi dispiace per voi meridionali, tutti quanti, sia da una parte che dall'altra.

Per tornare a parlare del FAS, signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la flessibilità nell'allocazione delle risorse che caratterizzano il Fondo per le aree sottoutilizzate consentono di impostare una politica nazionale regionale coerente con i principi e le regole di quella comunitaria e di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale. Non tutti, però, riconosciamo onestà intellettuale che la filosofia dell'azione del Fondo è mutata nel tempo e sulla base di precise leggi, a riprova che il FAS non è intoccabile. Anzi, per sua natura si presta ad una elasticità notevole. La finanziaria per il 2004, per esempio, ha rimodulato l'equilibrio tra incentivi e investimenti a favore di questi ultimi. La finanziaria per il 2005 ha invece modificato l'elenco degli strumenti alimentati con le risorse del FAS. La non lineare, seppur breve, storia del FAS mostra come di volta in volta sono stati aggiunti o modificati oneri e quantità di risorse. Quando poi si verifica che nel 2005 si sono riassegnati al FAS 526 milioni di euro per rinunce delle prenotazioni al credito d'imposta o addirittura 910 milioni sono rimasti inutilizzati per minori prenotazioni sulla base dell'articolo 7 della legge n. negli anni 2004-2006, il dubbio che parte delle risorse destinate non giungano ad alcun fine diventa realtà. Allora, come descrivere la diminuzione del FAS di 282 milioni di euro destinati nel 2006 a favore della Regione Sicilia per coprire spese già effettuate? O parlare di sottrazione di risorse per il Sud a proposito dell'utilizzo, nel 2008, di 450 milioni di euro del FAS per la crisi dei rifiuti in Campania e di 240 milioni di euro nel triennio per la crisi dei rifiuti in altre città del Mezzogiorno? degli 800 milioni che si destinano a Roma e Catania, in situazioni diverse di difficoltà, si può dire che non vengano concessi per superare difficoltà di aree del Centro-Sud?

nel tempo gli stanziamenti del Fondo rispetto alla finalità di ridurre il divario economico soprattutto in termini infrastrutturali e di rispettarne la proporzionale ripartizione tra le aree del Nord

al Sud. È interessante notare questo fastidio perché oggettivamente disvela un effetto speciale utilizzato durante le elezioni politiche, rivela un trucco (la parola mi sembra forte), quasi un inganno elettorale,

Visto che non è un problema di quantità, discutiamo della qualità. Restituite il maltolto! Ma è inutile affrontare questo tipo di argomentazioni, è inutile discutere

Vogliamo parlare di come vengono distribuite le pensioni in Italia? È inutile provare a spiegare che c'è un interesse complessivo del Paese, quello di affrontare in maniera

va considerato un altro effetto speciale: siamo nuovamente alla tecnica elettorale, il problema è diventato quello del funzionamento. Non sarà così. Senza risorse il Sud è destinato ad essere sempre più affossato. La questione è che il patto sociale, territoriale e politico che sostiene la maggioranza che ci governa si regge sulle spalle dei più deboli e quindi anche sul Sud. Anche per questo non si capirà lo spirito delle proposte avanzate dal PD che vanno nell'interesse complessivo del Paese e non solo di una sua parte.

la valorizzazione della classe dirigente meridionale e un maggiore investimento del Governo in termini di progetti e di servizi. Vi è una straordinaria occasione di rilancio dell'economia meridionale che deve andare di pari passo con il tema delle infrastrutture.

Ma la questione centrale, per agganciare il Sud al resto del Paese e all'Europa, è rappresentata da una priorità nell'attuale crisi economica internazionale: superare e ridurre il divario territoriale che storicamente divide il nostro Paese, il Nord dal Mezzogiorno. Lo dico da uomo del Sud che quotidianamente si impegna nella Regione di appartenenza, una delle Regioni più maltrattate del Paese: la Calabria.

oggi ammontano a 64 miliardi di euro, così come previsto dalla legge n. 296 del 2006, e per l'85 per cento sono in favore del Mezzogiorno, anche attraverso i cofinanziamenti dei programmi a valere sui fondi strutturali 2007-2013. Quindi, la crescita del Paese dipende anche dallo sviluppo del Meridione. In particolare, gli interventi strutturali devono avvenire secondo le procedure previste dagli accordi di programma quadro, con priorità per gli interventi nei settori della sicurezza, dei trasporti, della ricerca, dell'acqua e del rischio idrogeologico. Con la mozione che ci accingiamo ad approvare impegniamo il Governo a predisporre un provvedimento che, contemporaneamente al decollo del federalismo fiscale, agevoli anche fiscalmente le iniziative imprenditoriali del nostro Mezzogiorno. Questo Governo dovrà capire nei fatti che è necessario spostare il baricentro della politica a favore del Mezzogiorno, verso incentivi di carattere non discrezionale, al fine di ridurre i costi di transazione e di intermediazione che hanno finora ridotto l'efficacia delle misure adottate. In questa prospettiva occorre verificare la praticabilità di misure di vantaggio fiscale per l'iniziativa imprenditoriale nel Mezzogiorno, nonché puntare su una forma di contrattazione decentrata in grado di valorizzare le particolari condizioni vigenti nel Mezzogiorno e di favorire l'occupazione. Purtroppo, nel Sud il modello delle Regioni della sinistra è fallito perché in Campania, in Calabria, in Puglia non vi è stata attenzione dedicata ai territori, ma si sono formate oligarchie

per coprire le pagine vergognose sui rifiuti tossici e radioattivi. Devo pur dire però che quelle navi stanno là, cari amici e colleghi, da oltre vent'anni; non sono state

sanitaria, ad esempio. Nella nostra Regione accumuliamo un *deficit* storico di 2 miliardi e 300 milioni, pari a metà del *deficit* nazionale della sanità

fine al mancato rispetto della legge in quella Regione. Quando manca la certezza del diritto, nel Mezzogiorno manca anche la certezza della democrazia. Ecco perché, cari amici della sinistra, siamo d'accordo sui temi che voi sollevate, ma dovete anche essere d'accordo sulle vostre negligenze e colpe che si sono sono accumulate in questi anni nel Mezzogiorno d'Italia. Il ritardo del Sud dipende soprattutto da questa mancata capacità di organizzare i territori e di dare risposte concrete all'occupazione del Mezzogiorno. Ci assumeremo le nostre responsabilità, ma voi dovete avere il coraggio morale di fare altrettanto di dare la possibilità al Mezzogiorno di riscattarsi da antichi ed atavici ritardi, ma soprattutto di porre fine a queste sequele clientelari che avete messo su nel Mezzogiorno, in una sovrastruttura oligarchica che attraversa il potere vero delle Regioni, che spesso

Compagna, illustre meridionalista e uomo che vive i problemi del Sud, con convinzione, per porre fine allo stillicidio del Mezzogiorno, dando la possibilità a tutti di avere la speranza di un futuro migliore, che guarda alle nuove generazioni con più attenzione e che arresti

Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola per trattare un argomento così delicato e controverso, sul quale normalmente siamo abituati a dire o pensare che le colpe sono sempre degli altri. A mio avviso, se il Meridione si trova in queste contraddizioni ed è in ritardo di sviluppo, sicuramente dobbiamo chiederlo a noi stessi:

partendo anche da una fantomatica industrializzazione in un territorio sicuramente non vocato a queste finalità. Oggi, il riemergere del meridionalismo nel dibattito politico italiano è sicuramente un fatto estremamente importante,

sicuramente non hanno rappresentato una condizione per la crescita del Mezzogiorno. Oggi c'è molta insoddisfazione, vengono rivendicate ulteriori risorse dimenticando che nelle casse delle Regioni del Meridione ci sono un'infinità di finanziamenti che, se spesi bene, potrebbero effettivamente cambiare le infrastrutture del Mezzogiorno. Allora credo che bisognerebbe fare luce su questi ritardi, bisognerebbe capire perché ancora oggi le risorse vengano spese impropriamente e non

non viene coniugata con le esigenze del lavoro e dell'occupazione: i nostri giovani vengono spesso preparati per un lavoro che non esisterà mai.

parassiti che poi non sanno come organizzare la propria vita, credo che sia un grande errore che commettiamo nei confronti di quei giovani che sono alla ricerca di una di una prospettiva futura. Cosa significa oggi questa rivendicazione infinita di risorse? Quando nelle casse di una Regione ci sono ben 11 miliardi

perché noi dobbiamo individuare tutto ciò che può servire a creare le condizioni migliori per la crescita. È vero che noi siamo in un'area marginale rispetto ai grandi mercati del Nord e del centro Europa e che abbiamo un costo che è sicuramente più elevato rispetto al resto d'Italia. Pertanto, respingendo con forza l'idea delle gabbie salariali, che sarebbero un insulto al buonsenso, noi diciamo però che dobbiamo farci carico dei problemi riprendendo quello che era un grande progetto progetto di Berlusconi: il corridoio Berlino-Palermo va ripreso ed attuato quale elemento funzionale allo sviluppo del Meridione, così come il ponte sullo Stretto di Messina, di cui si parla da tanto tempo,

potesse costituire un'occasione importante ed interessante per una riflessione onesta sulla condizione del Mezzogiorno. invece con vero dispiacere che, valutando il dibattito che si è finora svolto, piuttosto che

il Senato si è voluto contraddistinguere - soprattutto dai banchi della maggioranza - per le tragiche assenze e per una supponenza culturale che è emersa negli interventi di alcuni colleghi. Voglio citare in particolare la collega Spadoni Urbani, che ha esplicitamente ritenuto di dover invitare - in maniera materna, devo non posso parlare di paternalismo - il Sud a rimboccarsi le maniche; ha ritenuto di dover affermare che il Sud non è capace di risolvere i propri problemi perché, è stato detto testualmente, «nel Sud albergano e vivono molti ignoranti».Ma questa affermazione - così come quelle che altri colleghi, in maniera meno evidente e più sfumata ma altrettanto grave, hanno ritenuto di dover proporre all'Aula - fa il paio con atteggiamenti di vera propria protervia istituzionale che uomini del Governo Berlusconi sovente hanno espresso. Cito per tutti l'ineffabile Brunetta che, dall'alto delle proprie valutazioni, potremmo dire, ha ritenuto di dover affermare che le donne e gli uomini della pubblica amministrazione del Sud valgono meno degli altri. Signor Presidente, cari colleghi, visto che il nostro Parlamento - ahinoi! - piuttosto che assolvere la propria funzione istituzionale

Cerchiamo di non perdere l'opportunità anche per esprimere a voce alta la nostra indignazione per il furto legalizzato che il Governo ha compiuto scientemente ai danni delle Regioni del Sud. I fondi per le aree sottoutilizzate, quelle poche decine di miliardi destinati al Sud, sono stati saccheggiati dal Governo: quasi la metà di quei fondi è stata utilizzata per altri scopi. Voglio citarne alcuni, che sono già stati evidenziati da altri colleghi: sanare i bilanci dei Comuni di Roma e Catania; trovare le coperture per il taglio che era stato promesso in campagna elettorale a proposito dell'ICI; coprire l'emergenza rifiuti; pagare il monopolio della Tirrenia.

dove, piuttosto che fotografare una situazione complessivamente critica di un'area che ha bisogno non di essere sfamata, ma sostenuta, si è pensato paternalisticamente di tirar fuori una ricetta che più o meno può essere rappresentata con il sistema del buffetto sulle guance, quasi come per dire: «State tranquilli perché, finché ci saremo noi, le cose funzioneranno».

alla quale, a dispetto delle notevoli frequentazioni del Premier in terra di Sardegna, è stata tolta - elenco soltanto qualche opera - l'opportunità di vedere il progetto sulla salute per il Mezzogiorno (189 milioni), il programma rete e mobilità per le strade (131, 125 e 500 milioni), la strada Olbia-Sassari, che è la vergogna dell'Italia. Signor Presidente, in questa strada in 14 anni sono morte 73 persone. La Regione e il Governo Prodi avevano trovato 500 milioni per realizzare la strada; il Governo Berlusconi ha tolto quei 500 milioni, perché ha ritenuto di doverli impiegare altrove. Mentre si commettono questi scippi e furti la gente continua a morire. Altri soldi sono stati tolti per le modifiche di Porto Torres, Sulcis, Ottana e Sant'Antioco, salvo poi aver visto il presidente Berlusconi in campagna elettorale, di fronte alle migliaia di lavoratori nel settore chimico che erano consapevoli di essere prossimi alla fame, prendere il telefono per chiamare in diretta l'amico Putin al quale, sempre con tono paternalistico, ha rappresentato una condizione che poi non è stata risolta. Colleghi, credo che il Senato si accinga accinga a perdere un'occasione importante per dare il proprio contributo ai problemi del Mezzogiorno. Non altrettanto farà il PD, che questi problemi li ha sempre vissuti e che li porterà avanti fino a quando non troveranno soluzione.

Sulla vicenda dei fondi FAS questo Esecutivo rivela la mancanza di una convincente strategia per risolvere l'attualissima questione meridionale. In questo ultimo anno il Governo ha utilizzato le risorse del FAS come un pozzo senza fondo, e ciò accade a discapito delle speranze del Mezzogiorno. Con l'abolizione dell'ICI per le case di lusso e la copertura degli scandalosi ammanchi e delle gravi situazioni debitorie di amministrazioni comunali di centrodestra avete dato la cifra del vostro impegno per il Mezzogiorno. Non ha stupito la stima della SVIMEZ che per il 2009 ha previsto una recessione al Sud dello 0,9 a fronte dello 0,6 nazionale. Nonostante tutto, il Governo pervicacemente in malafede ignora questa emergenza. I provvedimenti varati portano allo smantellamento dell'automatismo del credito d'imposta; si sono abbattuti gli investimenti produttivi e contestualmente non si è fatto nulla sul fronte dei consumi a tutela dei salari bassi. Il vento però sta cambiando: i cittadini del Sud e i siciliani stanno scoprendo sfortunatamente sulla loro pelle la catastrofica azione antimeridionalista del Governo Berlusconi. Tutto questo lo avete fatto senza il confronto con le Regioni. Siamo stanchi di un meridionalismo di facciata e del trasformarsi di colleghi meridionali in belle statuine, in "signor sì" silenti ed incapaci di indignarsi perché sono sempre sotto ricatto. Il centrosinistra aveva portato a 64 miliardi il FAS, implementando l'automatismo sul credito d'imposta per le imprese e ha sgravato dell'imposta sulla prima casa le famiglie povere. Senza il Meridione, l'economia e l'Italia non ripartono. Il Mezzogiorno sta pagando il prezzo più alto per le infrastrutture, essendo condannato a più alti costi energetici. Il Sud non può essere considerato un'inutile zavorra per il Paese: il Mezzogiorno e la Sicilia sono grandi opportunità a disposizione dell'intera Nazione per uscire da questa desertificazione dell'economia reale. La Sicilia è la piattaforma naturale nel Mediterraneo, può e deve divenire testa di ponte con i Paesi che si affacciano sul *Mare* *nostrum*, centro di stoccaggio per le autostrade del mare, ma anche terra e piattaforma di culture diverse, sede di un circolo virtuoso tra arte, cultura, natura, sole, mare, eccellenze e agricoltura. Abbiamo, invece, assistito ad un raggiro intollerabile. Dopo esser stato costretto a confermare i 27 miliardi stanziati dal Governo Prodi assegnati direttamente alle Regioni, il *dream* *team* berlusconianoha bocciato i piani attuativi determinando l'indisponibilità delle risorse per le Regioni e per il Sud. Nel caldo d'agosto il Premier, inseguito dalle cronache nazionali e internazionali, ha tirato fuori dal cilindro i soliti effetti speciali: la nuova Cassa per il Mezzogiorno, una nuova banca e un'Agenzia per il Sud. Il piano Marshall, così da lui definito, è stato subito azzerato dalle reprimende della Lega. Del corridoio Berlino-Palermo non si parla più; l'adeguamento della rete ferroviaria Palermo-Catania e Palermo-Messina è stato archiviato ed ai parlamentari siciliani del PdL è stato messo il bavaglio con le elargizioni a fondo perduto concesse alle amministrazioni a guida PdL di Catania (200 milioni), per i buchi di bilancio, e di Palermo, per la mala gestione dell'azienda dei rifiuti (150 milioni), che non basteranno a coprire i danni creati dall'allegra gestione, dalle assunzioni clientelari e dallo sperpero di risorse, anche con viaggi esotici

ma vi assicuro che non si sono fatti mancare niente: andavano lì per individuare possibili nuove attività che l'AMIA non avrebbe potuto avviare negli Emirati Arabi, essendo una società *in house*. Grazie ad un decreto, Berlusconi consente al sindaco Cammarata - coinvolto in uno *scoop* fatto emergere da «Striscia la Notizia», che ha creato indignazione tra i più - di raddoppiare l'addizionale IRPEF, in barba allo stesso Consiglio comunale, che per legge è preposto all'approvazione di una specifica delibera. Salutiamo positivamente, anche se non può consolarci, la scelta della magistratura di avviare processi contro la vicenda dell'AMIA e l'apertura di un fascicolo sulla vicenda della barca del sindaco di Palermo. Certo, è confortante la scelta di tutte le organizzazioni datoriali e dei lavoratori di ricorrere al TAR contro le nefaste scelte del Governo di centrodestra. E mentre il presidente Trichet conferma che la crisi non è finita e invita le banche a dare soldi alle imprese, gli imprenditori acquistano spazi televisivi e pagine di giornali e avviano uno sciopero della fame davanti alle banche per chiedere risposte concrete agli istituti di credito e allo stesso Premier. Si tratta di imprenditori che con difficoltà scelgono la strada della denuncia contro il *racket* e le estorsioni, mentre la presidente Marcegaglia chiede

ad Agrigento, il Presidente della scuola di calcio dedicava la vittoria ad un suo amico, ilboss di Palma di Montechiaro, arrestato in questi giorni. La cultura mafiosa ha ancora un forte *appeal*, ma diciamo che mentre con volontà, rigore e coraggio gli imprenditori denunciano gli estorsori, si incatenano e digiunano, il centrodestra, che ha importanti esponenti che considerano Mangano un eroe, vara lo scudo fiscale per far rientrare impunemente e nell'anonimato fondi che riposavano in paradisi fiscali, frutto di evasioni, di riciclaggio del denaro dei mafiosi, sporco del sangue di tante vittime della mafia. È questo il vostro impegno per il Mezzogiorno, ma fortunatamente anche in Sicilia comincia ad avanzare l'indignazione. Qualcuno ci ha chiamato farabutti: parlate con quel 30 per cento dei siciliani che vive sotto la soglia di povertà e cominciate a chiedere loro cosa pensano di voi, delle vostre false promesse e delle vostre bugie. Mandate in Sicilia (a Palermo e Catania,

e, se è coerente, chiederà scusa a quelli che chiama fannulloni. In ultimo, un augurio per il trentasettesimo compleanno del Premier, che oggi è in Abruzzo a consegnare nuove case ai terremotati: lo dica che gran parte delle risorse per la ricostruzione provengono dal Fondo per le aree sottosviluppate; almeno, signor Presidente, per il suo trentasettesimo compleanno, non dica bugie.

dovremmo evitare di trattare la questione del Mezzogiorno per farne un terreno di scontro tra opposte fazioni, tra coloro che si ergono a difensori del Mezzogiorno e quelli che invece, a sentire alcuni, lo dimenticherebbero, con le sue acute aspettative. Credo che nessuno debba fare torto ad un approccio che abbia il profilo di una sostanziale onestà di valutazione: a parte le cause storiche, la questione non è di oggi e ha radici antiche; c'è stato di mezzo un intervento straordinario, durato fino agli anni '80, ma che comunque ha fatto vivere un approccio sistemico nell'affrontare le problematiche dello sviluppo del Sud. Non dimentichiamo che nel periodo 1951-1973 il rapporto tra investimenti e PIL nel Sud era passato dal 17 al 33 per cento e che nel 1995 si era tornati al livello di investimenti del 1950; ciò per dire che la storia va vista nel suo insieme. Il merito di una logica di sistema nella programmazione degli interventi si è poi perso nella segmentazione Regione per Regione, dove la somma degli interventi non poteva fare, come non ha fatto, il Meridione come insieme. Il problema allora è l'ammontare delle risorse - che pure è un problema - oppure la modalità con cui queste si sono spese negli ultimi anni? Se si sommano tutte le risorse dell'ultimo ciclo comunitario 2000-2006 si arriva ad una cifra di 80 miliardi di euro, non poco. Di questi, al netto dei cosiddetti progetti sponda - per capirci, quella invenzione tecnica che ha consentito la rendicontazione di spese estranee alla originaria programmazione - ne sono stati spesi solo 43 miliardi, con una percentuale del 53 A questa valutazione quantitativa, per niente lusinghiera, si aggiunge una valutazione qualitativa altrettanto insufficiente, se al compimento dei programmi è difficile riscontrare nelle Regioni dell'Obiettivo 1 il raggiungimento di quegli obiettivi di rafforzamento produttivo, infrastrutturale e di avvicinamento Allora, nessuno di noi deve avere questa amnesia, perché qui si giudicano responsabilità trasversali. Chi ha guidato in questi anni, e per lungo tempo, Regioni come la Calabria, la Puglia, la Campania, la mia Basilicata ha egualmente avuto responsabilità di Governo sul piano nazionale. nazionale. Forse è più utile guardare ai problemi e alle criticità che si sommano nel Mezzogiorno piuttosto che strumentalizzarli, senza proposte che siano coerenti con le politiche nazionali, con i vincoli di finanza pubblica e con gli scenari globali che come Paese abbiamo davanti. Cosa dobbiamo fare per arginare il fronte polemico dell'attuale opposizione a proposito del taglio dei fondi FAS? Ricordare che il Governo Prodi fece altrettanto con tre atti della manovra finanziaria del 2008 attingendo anch'esso al FAS? Diciamo la verità, in questi anni tali fondi si sono trasformati in una sorta di polmone finanziario, ridotto o ricostituito a secondo delle necessità della effettiva erogazione della spesa. Dunque, il problema non sono i fondi FAS, ma piuttosto il destino e l'impatto che i programmi di spesa hanno avuto e avranno nelle aree del Mezzogiorno. Un giudizio che non è estetico né accademico, ma che richiama l'assunzione di atti di governo e di coordinamento all'inizio di un nuovo ciclo di spesa che per molte Regioni del Sud potrebbe essere l'ultimo con il sostegno europeo. le risorse che abbiamo davanti sono importanti: si stimano almeno 60 miliardi di euro tra risorse comunitarie e risorse nazionali. Esiste quindi una realtà concreta per far fronte a questa esigenza. Diceva il nostro Capogruppo vicario, senatore Quagliariello, che se i capitali non ci sono ma creiamo le condizioni attrattive, i capitali alla ricerca di redditività arrivano. Per questo dobbiamo incrociare politiche regionali e politiche nazionali, per superare i fattori negativi che oggi frenano il Sud: si chiamano infrastrutture, capitale umano, nuovi incentivi all'intrapresa. Il Sud è una grande occasione per l'intero Paese, lo sanno anche gli amici della Lega,

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, sono state richiamate ripetutamente in questo dibattito le cifre e i numerosi decreti legge con cui di volta in volta avete attinto - mi riferisco al Governo - ai fondi FAS per sostenere spese del tutto estranee alle finalità di tale Fondo: una lunga serie di atti e provvedimenti che hanno rappresentato un duro colpo alle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno.

il finanziamento degli interventi anticrisi, al contrario di altri Paesi, è stato assicurato principalmente da interventi di riallocazione e rimodulazione delle risorse pluriennali destinate, in larga misura, a interventi infrastrutturali. Infatti, gran parte delle maggiori spese sono state compensate mediante tagli, riprogrammazioni e riallocazioni delle risorse nazionali finalizzate soprattutto allo sviluppo del Mezzogiorno, presenti nel Fondo per Ed ancora, si legge nel Rapporto che nel corso del 2008 e nei primi sei mesi del 2009 il legislatore è intervenuto con rilevanti utilizzi della dotazione FAS per impieghi sovente non coerenti con le finalità proprie del Fondo.

Avete motivato tali scelte sostenendo che bisognava rispondere alle emergenze del Paese e che si trattava di utilizzare risorse che tanto si sprecavano o che restavano inutilizzate: avete fatto vostro, insomma, un pregiudizio prima culturale che politico, che spesso si è ascoltato nelle feste padane o si è letto su certa stampa nazionale e che Tremonti ha, con più eleganza, fatto proprio: l'idea del Sud sprecone ed incapace a cui bisognava fargliela pagare, concentrando a Roma il luogo delle scelte e sottraendolo alle Regioni. Un'idea che si fa strada, che tende a generalizzare il giudizio negativo su errori, inefficienze, sprechi che nel Mezzogiorno certo ci sono stati e che sono davvero in pochi oggi a non vedere o a tentare di nascondere: una capacità di analisi che è e deve essere altra cosa dal giudizio tranciante su intere classi dirigenti o su intere Regioni e che serve solo a dare fiato a due considerazioni: che non ci sia più una questione meridionale e che le risorse è meglio che le gestisca qualcun altro. Ed è paradossale che tale politica si affermasse nei mesi scorsi proprio mentre il Parlamento nazionale - lo direi al ministro Tremonti se fosse presente, lo dico ai colleghi della Lega approvava, con il nostro contributo essenziale, la legge quadro sul federalismo fiscale, esaltando, quindi, il ruolo delle autonomie locali. E come dimenticare che con uno dei tanti decreti-legge avete scelto di svuotare il credito d'imposta per gli investimenti delle imprese meridionali? Uno strumento che il centrosinistra aveva rafforzato rendendo automatici i contributi e che oggi viene in qualche modo svuotato. E se gli atti parlamentari hanno ancora un senso in questo Paese, come dimenticare ancora programmazione economico-finanziaria 2010-2013, lo strumento più importante di programmazione economica e finanziaria, in cui non c'è una parola rivolta al Mezzogiorno, che viene letteralmente espulso

della sua fertile fantasia ieri a Napoli su proposte che farebbe meglio ad avanzare qui, in Parlamento, magari presenziando a questo dibattito. E se queste proposte sono la realizzazione concreta degli strabilianti annunci di prima dell'estate del presidente Berlusconi di improbabili piani straordinari per il Mezzogiorno, è il caso di dire che la montagna ha partorito il topolino. Ed allora, continuiamo a pensare che ci sia ancora in questo nostro Paese una grande questione irrisolta, quella meridionale, che oggi va assunta e declinata certamente in forme nuove: a cominciare dall'analisi, che se attenta ed oggettiva, ci consegna grandi problemi, ma anche veri e propri punti di eccellenza, nell'impresa come nella ricerca, nella formazione di eccellenza come nelle buone prassi amministrative, nella liberazione dalle mafie come nella cultura e nei saperi. Penso a quell'Arcipelago dei saperi che nei prossimi giorni a Napoli riunirà scienziati e ricercatori del Mezzogiorno e di tutto il mondo. Una questione che ha bisogno non solo, ma senza dubbio e senza ipocrisie, anche di risorse: soprattutto del rispetto, dopo la cessazione dell'intervento straordinario, di quell'impegno, spesso tradito, di garantire risorse aggiuntive di origine comunitaria ai trasferimenti ordinari interni. Se il Mezzogiorno, insomma, è il problema dell'Italia, è altrettanto vero che solo la soluzione di tale problema - di una parte del Paese così grande con gravi *deficit* di sviluppo - può aiutare l'Italia intera a tornare ad essere competitiva sulla scena internazionale e a superare la stessa grave crisi in atto. Per dirla con le parole dell'ultimo lavoro di uno dei pensatori più moderni ed attenti del Mezzogiorno, Franco Cassano, l'autore di quel pensiero meridiano che quasi venti anni fa esaltava il paradigma dell'autonomia del Sud come soggetto, oggi, signor Presidente, colleghi, «occorrono politiche nazionali ed internazionali: per togliere il Mezzogiorno dalla sua dimensione periferica bisogna pensare in grande».

su cui la retorica sembra aver sostituito la politica e la volontà concreta di aprire una pagina nuova». Noi abbiamo bisogno di pagine nuove.

È come se i fondi per le aree sottoutilizzate li avesse inventati Berlusconi e poi non li utilizzasse, o meglio, li utilizzasse per altre cose, come dice l'opposizione. Nessuno, Nessuno, da oggi pomeriggio in poi, ha fatto una riflessione sul modo in cui questi fondi sono stati utilizzati negli anni passati, sulla qualità della spesa degli stessi fondi, che hanno comunque testimoniato e sottolineato un dato, che nel Mezzogiorno d'Italia non sono mancate le risorse, ma la capacità di dare loro una finalizzazione produttiva e virtuosa. Credo che una classe dirigente responsabile, una istituzione e i parlamentari che siedono nel Senato debbano partire da questo dato per fare una riflessione sull'utilizzo dei fondi per le aree sottoutilizzate.

tutti alla ricerca di un responsabile di turno per allontanare da sé stessi eventuali responsabilità, fino ad arrivare,

Ogni occasione della politica, a seconda del modo in cui la si legge, è una pantomima, un teatrino, una sceneggiata o una farsa. Basta che ognuno si regoli per dargli il significato che più calza nel momento in cui vuole costruire un discorso per sottolineare per sottolineare il dato negativo di un'iniziativa rispetto ai dati positivi che da questa emergono. Ripeto, c'è un problema sulla qualità dell'utilizzo delle risorse. Con grande chiarezza - poi veniamo anche alla sceneggiata, collega Armato

soprattutto la responsabilità, di spendere questi fondi, non solo quelli del FAS, ma anche gli altri, non hanno avuto grande capacità di programmazione per fare sistema dall'utilizzo di questi fondi. È un dato credo incontestabile, che sta sotto gli occhi di tutti quanti. Non si può pensare di fare un ragionamento

C'è anche un'altra questione che si inserisce nel dibattito in atto: poteva o doveva il Governo utilizzare al meglio le risorse disponibili per fare meno danni possibili all'economia reale e quindi mettere in moto un percorso per superare in maniera

l'utilizzo virtuoso dei fondi e la responsabilità del Governo (di qualsiasi Governo) di utilizzare le risorse disponibili per superare la crisi nel modo in cui tutti noi abbiamo visto.

Siamo alla tragedia ed è la tragedia che viene consegnata al Paese.

se con dolore (perché non dirlo) li ho abbandonati e non certamente con imbarazzo sono qui oggi a difendere le ragioni del Mezzogiorno

ma partito per il Sud, ovvero per affrontare una questione rimasta assolutamente irrisolta nell'arco di tanti anni.

si aspetta che, contestualmente alle tematiche del federalismo, che sono giuste e rispetto alle quali in termini di responsabilità non intendiamo minimamente tirarci indietro,

Non è un favore che si fa al Mezzogiorno se si interviene con fondi aggiuntivi! È un dovere di uno Stato che, attraverso il suo Governo, ha partecipato ad una contrattazione in sede comunitaria,

per un territorio che è ancora in ritardo di sviluppo e che, per affrontare il federalismo, deve essere messo alla pari con gli altri territori.

che pure si sarebbe potuto condividere. Allora, Presidente, credo che non si stia chiedendo niente di più che l'affermazione di un diritto, rispetto a risorse

di sinistra, eppure i fondi comunitari non sono stati tutti utilizzati. Né è lecito a nessuno confondere i fondi strutturali con i fondi per le aree sottoutilizzate: un minimo

se l'impianto è quello di creare risorse che determinino formule di cofinanziamento, è chiaro ed evidente che la programmazione 2007-2013

che chi non è riuscito a fare determinate cose in cinque anni difficilmente riuscirà a farle in un anno. Allora è evidente che anche in questo caso si vogliono sottrarre ulteriori risorse al Mezzogiorno d'Italia essere libera di poter dire finalmente queste cose, che invano ho tentato di far comprendere a qualcuno nel tempo.

la mozione presentata dal Gruppo PDL fa a mio avviso giustizia delle strumentalizzazioni che in questi mesi sono state messe in atto dalle opposizioni, chiarendo in modo inequivocabile la posizione del PDL non solo sulla vicenda del Fondo per le aree sottoutilizzate, ma più in generale sui problemi di sviluppo del Mezzogiorno e dell'intero Paese. Quello che è necessario sottolineare a corredo della nostra mozione, è l'approccio operativo alla questione dello sviluppo che intendiamo sostenere: nessuna tentazione di contrapposizione tra Nord e Sud, ma piena consapevolezza che federalismo fiscale e agevolazioni fiscali per le iniziative imprenditoriali nel Mezzogiorno rappresentano due facce dell'unica medaglia dello sviluppo nazionale. In questo senso l'impegno per la conferma delle percentuali di riparto dei fondi tra Centro, Nord e Sud può essere l'occasione per dismettere una polemica sterile e vana intorno alla presunta vocazione nordista del Governo e per concentrare le attenzioni su quello che è necessario fare per superare la scarsa competitività dei territori meridionali. Tuttavia, è anche necessario ribadire - al di là delle contingenze, spesso strumentali, del dibattito politico che la questione meridionale è una questione nazionale e, come tale, impone da un lato l'assunzione di provvedimenti urgenti, come quelli proposti dalla nostra mozione, ma dall'altro rende urgente anche un ripensamento generale delle modalità di approccio e di intervento pubblico nel Mezzogiorno d'Italia. Il problema del riparto dei fondi FAS ha dato nei mesi scorsi l'impressione, profondamente sbagliata, di un Sud che rappresenta una "voragine" del Paese, nella quale vengono dilapidati ingenti capitali senza alcuna produttività. Questa vecchia immagine del Sud piagnone e parassita deve essere smentita innanzi tutto dalle classi dirigenti meridionali, che sono chiamate ad uno sforzo straordinario sulla stessa idea di futuro dei propri territori. Questa nuova idea di futuro del Mezzogiorno d'Italia non può che essere incentrata sulle grandi priorità che minano alla base la sua competitività: la sicurezza pubblica e la realizzazione di un clima di legalità e trasparenza che favorisca lo sviluppo di investimenti e la valorizzazione dei territori; il rafforzamento dell'attrattività dei territori, attraverso adeguati interventi di dotazione infrastrutturale e di protezione e capitalizzazione delle risorse ambientali; lo sviluppo dell'economia della conoscenza e dell'innovazione che punti sulla valorizzazione del capitale umano, che è la vera ricchezza produttiva del Sud. In questo sforzo di ammodernamento e rilancio del Mezzogiorno, l'azione del Governo centrale è certamente fondamentale. Ma ancora una volta non sarà sufficiente se questi interventi non avranno il supporto, la condivisione ed il coerente sviluppo locale da parte delle classi dirigenti meridionali, alle quali viene richiesto - *hic et nunc* - questo impegno straordinario. La lezione che viene dal contesto economico internazionale, caratterizzato dalla continua crescita della concorrenza dei Paesi emergenti, chiama i territori meridionali a sostenere azioni di innovazione a sostegno del proprio tessuto produttivo e a ripensare le strategie legate agli obiettivi di competitività dei sistemi economici territoriali. La concorrenza tra imprese si va trasformando sempre più in concorrenza tra aree. Ciò determina la necessità di accrescere la *performance* di tutti quei fattori esterni alle aziende che contribuiscono a favorire l'innovazione e più in generale i processi di rafforzamento del sistema economico nel suo complesso. Così si sta rivelando fondamentale la prestazione istituzionale locale, intesa come abilità dei governi locali di usare in maniera efficiente ed efficace le risorse a disposizione per lo sviluppo delle economie territoriali. Ecco perché lo sviluppo del Sud è un impegno che coinvolge tutti: il Governo dovrà sicuramente fare la sua parte, ed il PdL è pronto a sostenerne l'azione di intervento immediato e concreto, ma i governi regionali dovranno concretamente dimostrare, attraverso i rispettivi Piani attuativi regionali, di tenere ben presente, da un lato il contesto di competizione nazionale ed internazionale nel quale operano, e dall'altro la necessità di assicurare la coerenza programmatica tra disegno nazionale e contesto territoriale; l'integrazione finanziaria tra risorse comunitarie e risorse nazionali del FAS; la reale addizionalità di tali risorse rispetto ai fondi ordinari. Sarà dunque un banco di prova per tutti! La speranza è quella di inaugurare una strategia unitaria e convergente di inaugurare una strategia unitaria e convergente tra Governo e Regioni per assicurare un livello di concentrazione degli interventi e delle risorse che segni la svolta definitiva nella dimensione territoriale dello sviluppo meridionale. Signora Presidente, colleghi senatori, prima dell'estate, insieme ai colleghi del Movimento per le Autonomie, abbiamo presentato una mozione che aveva ad oggetto un tema specifico, cioè l'utilizzo dei Fondi per le aree sottoutilizzate, con particolare riferimento con particolare riferimento alla questione della quota regionale di questi fondi, perché *l'impasse* che il Governo aveva segnato al riguardo aveva messo in ginocchio l'attività di programmazione delle Regioni in settori strategici e importanti per lo sviluppo di quelle comunità. Da qui si è sviluppato un dibattito surreale, a volte anche un po' ridicolo - mi si passi il termine - che ha avuto anche la presunzione di evocare partiti e così In realtà, la piccola, grande vicenda dei fondi FAS è la metafora della crisi di questa maggioranza di Governo; sotterranea ma profonda, che sta rendendo di fatto ingovernabile parecchie Regioni del nostro Paese. Paese. Non voglio assolutamente - perché non è questo il tema - entrare nel merito di tali questioni, ma c'è sembrato giusto ampliare il dibattito sul Mezzogiorno perché il problema reale è tentare di fare un'operazione verità sulle questioni che riguardano il Sud del nostro Paese con riferimento alle politiche nazionali, ma anche alle politiche delle istituzioni locali che concorrono oggi più di ieri a determinare gli indirizzi di sviluppo dei territori. Ci è sembrato quindi opportuno presentare mozioni più ampie che non fossero circoscritte solo alla questione dell'utilizzo dei fondi FAS, su cui però ovviamente ci intratterremo. Credo però che questo dibattito, signora Presidente, rischia di essere l'ennesima occasione mancata. Lo dico questa volta con polemica nei confronti del Governo: con tutto il rispetto per il signor Sottosegretario qui presente, credo sia scorretta l'assenza del ministro Tremonti in quest'Aula se, come i colleghi di maggioranza hanno detto, questo dibattito è importante,

Questa assenza non è casuale. È legata anche alla circostanza di questo balletto cui abbiamo assistito negli scorsi giorni in ordine alla mozione congiunta che i colleghi del Popolo della Libertà avrebbero dovuto sottoscrivere con i colleghi della Lega. Poiché non vi è traccia di una firma dei colleghi della Lega sulla mozione del Popolo della Libertà devo ritenere che non vi sia una visione comune della maggioranza e di questo Governo sui problemi del Mezzogiorno e devo ritenere che l'assenza del Ministro dell'economia, del Ministro per lo sviluppo economico e del Sottosegretario con delega allo sviluppo e alla coesione sociale non sia casuale ma sia dettata dall'assoluta impossibilità da parte di questo Governo di esprimere un'opinione - non un fatto concreto - identica su un tema così importante e delicato per l'intero Paese, non solo per il Mezzogiorno d'Italia. Devo aggiungere, signora Presidente, che è evidente che sia così perché il ministro Calderoli, che notoriamente ha la delega sul Mezzogiorno, ha dichiarato che l'unica ricetta per il Sud è il federalismo fiscale. fiscale. È chiaro ed evidente che, rispetto ad altre opinioni autorevoli esistenti in questa maggioranza, non vi può essere un'unità di intenti né una coesione del Governo e di questa maggioranza su questo tema. Non può esservi, perché è lì il vero problema. A me dispiace dover tornare su questo argomento, a rischio di essere noioso, ma la madre di tutte le questioni è il federalismo fiscale o, meglio, quella somma di due disastri rappresentati dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione,

erogazione, di controllo e di gestione della spesa pubblica. Ciò è tanto vero che oggi il ministro Tremonti ha dichiarato, in un comunicato alle agenzie

della spesa e della finanza pubblica in settori delicati e strategici per il nostro Paese, come la sanità, le professioni, il turismo e il settore dei trasporti. Tutto questo trova il marchio finale nella legge sul federalismo fiscale che, peraltro, in quella famosa norma riguardante la perequazione infrastrutturale, prevede una cabina di regia che è già

voi lo avete votato, insieme - lo dico senza polemiche - anche ai colleghi del Partito Democratico, e questa è la ragione fondamentale per la quale oggi qui si discute non di politiche nazionali attinenti ad aree diverse del territorio, ma ad una contrattazione sulle richieste di risorse che pezzi di territorio avanzano accampando pretese di natura politica. Questo è il tema e lo sfondo sul quale costruiamo e innestiamo questo surreale dibattito sul Mezzogiorno. In questo contesto, signora Presidente, è chiaro che anche le tre idee forti del ministro Tremonti

o una struttura pubblica? Si possono creare istituti di credito pubblico? È un sistema di coordinamento di piccole banche e istituti di credito? Di cosa stiamo parlando? Cosa è questo oggetto misterioso? Quando lo apprenderemo e sapremo cos'è, allora saremo anche nelle condizioni di capire

parla poi della defiscalizzazione, in sostituzione della fiscalità di vantaggio, dei depositi di chi mette i propri risparmi in banche del Sud.

rientrare somme della cui provenienza lecita tutti dubitiamo e tutti siamo preoccupati, visto che, con buona pace del Ministero dell'economia, la normativa antiriciclaggio non è superabile. A prescindere da questo, comunque, non vorrei che finisse come la cosiddetta

che dovevano essere utilizzati per spese infrastrutturali, cioè per investimenti che avessero effetti positivi nel medio e lungo periodo, per affrontare la crisi in maniera congiunturale.

ha fatto e ciò significa che purtroppo questa è la verità e di questo dobbiamo prendere atto

signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, i fatti messi in rilievo nella mozione presentata dal Gruppo dell'Italia dei Valori - la sistematica ed inarrestata sottrazione dei fondi per le aree sottoutilizzate a favore di finalità estranee alla natura di tali fondi - ha cause ed origini lontane. Nel 2004, commentando la recente introduzione del Fondo per le aree sotto-utilizzate, la SVIMEZ, nel suo rapporto annuale, scriveva: «Con la legge finanziaria per il 2003 le risorse aggiuntive nazionali a favore delle ex aree depresse sono state riorganizzate e concentrate nel Fondo aree sottoutilizzate. L'innovazione introdotta permette di collocare il CIPE quale luogo di indirizzo strategico unitario delle politiche di riequilibrio territoriale. Le procedure di trasferimento e di utilizzo delle risorse finanziarie presentano, però, ancora limiti e lati oscuri, che incidono, in prospettiva, sull'entità della spesa per investimenti per il Mezzogiorno. Tali procedure sono caratterizzate da forti elementi centralistici nell'assegnazione delle risorse e da potenziali conflitti tra Governo centrale e governi locali». Quanto previsto dalla SVIMEZ è quello che puntualmente si è realizzato: un Governo centrale fortemente condizionato da istanze antimeridionalistiche ha approfittato di un meccanismo debole e ciò ha provocato aspri conflitti con le Regioni ed il risorgere di sentimenti da tempo sepolti. Il tema che si pone è allora duplice, signora Presidente: da un lato sapere cosa è successo ed impegnare il Governo a ricondurre il FAS, nella quantità e nella qualità delle risorse, alle originarie finalità, dall'altro avviare una profonda riflessione su procedure di allocazione delle risorse che hanno consentito, di fatto, al FAS, di funzionare come bancomat per far fronte a esigenze ordinarie, anche di altre aree del Paese. Si può quantificare in oltre 18 miliardi di euro il totale delle riduzioni operate sul FAS tra il 2008 ed il 2009, somma a cui vanno aggiunti tra i 2.000 ed i 4.000 milioni per il terremoto in Abruzzo. La quasi totalità di queste somme sono state prelevate con decreto-legge. Va sottolineato non solo il prelievo dal FAS o l'utilizzo del FAS per finanziare spese in aree non sottoutilizzate, ma anche la tendenza all'impiego, nelle aree sottoutilizzate, a scopo sostitutivo e non aggiuntivo. A tal proposito occorre ricordare che il requisito della aggiuntività del FAS non è frutto di autonome scelte di politica economica nazionale, e come tale emendabile, ma è diretta conseguenza della riforma della politica di coesione comunitaria, che ha comportato l'unificazione della programmazione della politica regionale comunitaria, finanziata dai fondi strutturali, con quella nazionale. In altre parole, l'utilizzo ordinario di tali risorse straordinarie nazionali rischia di farci perdere consistenti risorse comunitarie. Altro tema messo in evidenza dalla nostra mozione riguarda la progressiva riduzione delle risorse economiche a disposizione di tutti gli enti locali: una situazione che va aggravandosi di anno in anno, in un processo che costringe Regioni, Province e Comuni a sopprimere servizi essenziali. Tali scelte ledono lo spirito del Titolo V della Costituzione e, specificamente, l'articolo 119 che - pur richiedendo per la sua puntuale applicazione appositi provvedimenti legislativi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, oltre che di istituzione del fondo perequativo fissa princìpi precisi, immediatamente vincolanti. Nel complesso quadro di difficoltà economico-finanziaria, l'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili, adottata con il decreto-legge

preoccupazione per l'assenza di un disegno organico di definizione del finanziamento locale e di misure indirizzate a sostenere la competitività e lo sviluppo, oltre che per la certezza di dover ridurre o sopprimere, per l'esiguità di risorse disponibili, dei servizi essenziali. Ieri il ministro Tremonti a Napoli ha parlato di un piano per il rilancio del Mezzogiorno; in particolare, ha suggerito di concentrare le risorse dello Stato sulle grandi opere pubbliche e di evitare i microinvestimenti. La speranza allora è quella di non trovarci più di fronte a ciò che è accaduto lo scorso anno quando il CIPE, in data 30 settembre 2008, ha assegnato, a fondo perduto, ai Comuni di Catania e di Roma rispettivamente 140 e 500 milioni di euro, per far fronte all'emergenza finanziaria dei due enti, coprendo tale spesa a valere sulle risorse FAS. Particolarmente allarmante risulta essere, a nostro avviso, il meccanismo di assegnazione dei citati contributi, le cui risorse finanziarie vengono individuate a valere sul Fondo statale per le aree svantaggiate, a sua volta fortemente ridotto da 64 a 57 miliardi di euro, dal decreto-legge

La delibera CIPE in oggetto, tuttavia, non è andata ad incidere su questa quota di risorse, bensì ha riguardato le «riserve di programmazione». Appare immediatamente evidente come, a fronte di oneri di natura corrente, le coperture siano individuate in risorse in conto capitale a valere sul FAS, il cui utilizzo risulta quindi strumentale ad un indebolimento e superamento del vincolo contabile, che non consente di coprire spese correnti con spese in conto capitale perché si verificherebbe una dequalificazione della spesa. Con la delibera del 30 settembre 2008 il CIPE ha assegnato formalmente i fondi ad un lungo elenco di piccole opere pubbliche, finalizzando così, nel rispetto delle regole di contabilità, risorse in conto capitale ad interventi infrastrutturali; tuttavia, i fondi assegnati dal CIPE al Comune di Catania serviranno nell'immediato a coprire fabbisogni di cassa più urgenti, quali il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici e dei fornitori, vista la situazione di dissesto finanziario dell'amministrazione etnea. Il Fondo aree sottoutilizzate costituisce dal 2003 lo strumento generale di governo della nuova politica regionale nazionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate. La strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la flessibilità nell'allocazione delle risorse, che caratterizzano tale Fondo, Fondo, consentono di impostare una politica nazionale e regionale coerente con i princìpi e con le regole comunitarie e di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale, solo e soltanto in conto capitale. Tale condizione risulta peraltro essenziale per soddisfare il principio di addizionalità, scaturente dagli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea. Nella vicenda che ho voluto richiamare c'è da fare un'ulteriore specificazione. Il finanziamento volto

il Mezzogiorno continua ad essere pesantemente colpito. Non vi è traccia nel disegno di legge finanziaria per il 2010 appena varato dal Consiglio dei Ministri del grande piano per il Mezzogiorno annunciato dal Governo. Rimangono sulla carta unicamente il taglio di quasi 2 miliardi di euro alle risorse dedicate alle infrastrutture di Sicilia e Calabria per coprire il taglio dell'ICI e, ancora, la revoca della programmazione dei Fondi per le aree sottoutilizzate, che hanno contribuito a passare da un quadro di certezza ad uno di totale incertezza. Gli interventi fino

alla Lega Nord preme che nel Mezzogiorno ci sia un'economia di mercato, che viva sul mercato e di mercato. Più che di quantità di risorse, a me sarebbe piaciuto fare un dibattito su come vengono spese le risorse e, quindi, sui fattori scarsi della competitività del Mezzogiorno e su come un investimento può rimediare in tal senso. Facciamo qualche esempio.

Ciò che non ci stupisce è che la causa principale della scarsa competitività del sistema Paese Italia non è, come potrebbe pensare il cittadino della strada, l'importo della tassazione (che sta al secondo posto), secondo posto), ma l'inefficienza della macchina della burocrazia. Per gli imprenditori di questo Paese il fardello più grosso è l'inefficienza della burocrazia.

le università meridionali, salvo qualche rara eccezione, sono sotto la media e non accedono ai fondi premiali. Tutti insieme dobbiamo, quindi, porci una riflessione su questi temi perché una classe dirigente non si forma abbassando il livello di selezione dell'istruzione scolastica, semmai facendo il contrario e ponendosi degli obiettivi più forti sulla formazione non solo professionale, ma soprattutto universitaria e su quella

cambiare argomento: anche qui, non bastano i luoghi comuni, perché sappiamo tutti che nel Meridione d'Italia vi sono molti posti bellissimi;

probabilmente le cose sarebbero diverse e il turismo avrebbe anche la possibilità di decollare più velocemente. E ancora, in materia di rifiuti è evidente che le cose non vanno bene e c'è poco da dire, perché lo sappiamo tutti: mancano soprattutto gli impianti,

del lavoro nero, come dimostrano i dati sull'evasione fiscale. Infatti, nel momento in cui in Calabria ogni 100 euro dichiarati se ne spendono 150,

risorse, è questo: vorremmo davvero sentire la ricetta da parte di tutti per portare nel Meridione più lavoro e meno posti di lavoro, più responsabilità e buona amministrazione.Questo è l'intendimento della Lega Nord*.

al senatore Garavaglia gli interventi di questo Governo a favore di singole città disastrate del Sud per smentirlo già in partenza, ma non è questo lo spirito del mio intervento. Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio raccogliere in pieno

perché ognuno le individua negli altri. Se questo è il modo con cui ci accostiamo al problema del Mezzogiorno non possiamo che denunciare il fallimento del Parlamento e delle forze politiche:

alle politiche carenti del Governo nazionale. Io non starò a ripetere il lungo elenco di inadempienze. Il problema vero sapete qual è? Lo dite voi in questa mozione, quando dite esplicitamente di impegnare il Governo a predisporre un piano per il Mezzogiorno: implicitamente ammettete che questo Governo non ha mai avuto un'idea sul Mezzogiorno. Siete venuti in Aula con il vostro programma, avete per due volte approvato un Documento di programmazione economico-finanziaria e oggi implicitamente ammettete l'assoluto vuoto di pensiero e di pianificazione sulla questione meridionale quando dite:

manca nel testo qualsiasi riferimento all'Agenzia, alla Banca del Sud. L'ho fatto notare amabilmente al senatore Compagna, il quale altrettanto amabilmente ha citato l'intervista che Tremonti ha rilasciato a «Il Mattino».

voi chiedete che ci sia un piano organico del Governo, possiamo noi chiedere al Governo di venire in Aula tra un mese o due per

a deporre ogni e qualsiasi argomento di natura polemica, che pure è facile adottare. Ci impegniamo a lavorare serenamente su una questione che è nazionale, purché il Governo non chiediamo molto - si presenti in quest'Aula e ci proponga, anche in modo aperto, un progetto organico sul Mezzogiorno. Noi siamo pronti a collaborare. una nuova finestra") *(PdL)*. Signora Presidente, sono d'accordo con la premessa e con la conclusione del senatore Procacci, anche se poi non si è saputo sottrarre neanche lui alla tentazione della polemica e dell'accusa alle spalle. Noi proponiamo che il Governo si impegni a predisporre un piano per il Mezzogiorno, e questa mi sembra una richiesta assolutamente dovuta. Mi sembra infatti che ciò rientri nella logica di una programmazione

sostenere che si risolve il problema con una delibera di assegnazione ad una Regione piuttosto che ad un'altra di cifre delle quali non conosciamo neanche la destinazione. La nostra mozione è molto semplice: non solo impegna il Governo a predisporre un Piano per il Mezzogiorno che, naturalmente, non potrà non passare per il dibattito nelle Aule parlamentari (spero anch'io che sia un dibattito di ben altri contenuti rispetto a quello di quasi

Il divario in termini di infrastrutture è palese, è dinanzi agli occhi di tutti, basta percorrere le strade di questa Nazione per capire che esiste un divario infrastrutturale tra Nord e Sud. è divario anche nei termini della considerazione che si ha dell'economia del Sud rispetto ad economie di altre zone non solo dell'Italia, ma dell'intera Europa. Il Sud è sempre stato considerato e utilizzato come momento è giusto che questa lontananza dai mercati, dal punto di vista delle produzioni del Sud, venga compensata con politiche non assistenziali, ma di intervento. La fiscalità di vantaggio sicuramente è un metodo per compensare il divario dovuto alla lontananza dai mercati, ma così dovrebbe essere anche la rivalutazione delle potenzialità del Mezzogiorno d'Italia. Penso, ad esempio, alla centralità mediterranea. Se interpretiamo la posizione del Mezzogiorno d'Italia non come periferia dell'impero, ma come luogo di centralità mediterranea

internazionali che riguardano il nostro Paese e il Mediterraneo si possano celebrare nei siti che la geografia, la storia e la cultura del nostro Paese indicano, cioè quelli del Sud d'Italia. Di conseguenza, il problema della competenza a destinare le somme è molto sterile riguardo a questo dibattito, perché sappiamo benissimo che chi oggi critica il centralismo nazionale, quando poi scende nelle sue realtà locali, si pone come centralismo regionale contro gli enti locali, a danno delle stesse istanze dei territori. Dunque, occorre una programmazione generale. Del resto, lo prevede la legge: i fondi FAS si utilizzano con accordi di programma. Gli accordi di programma sono intese tra il livello nazionale che eroga le somme e il livello regionale che fa la proposta di utilizzo: insieme si decide come utilizzarli. È la legge che lo dice; quindi, nulla di scandaloso se si chiede al Governo di predisporre un piano; nulla di scandaloso se si chiede alle Regioni di rinunciare a gelosie di competenze, che molto spesso mascherano incapacità o volontà di utilizzazione delle somme al di fuori dei canoni previsti dalla legge; nulla di scandaloso, quindi, se anche nella programmazione dei fondi europei si trovi una *liaison* con l'utilizzazione dei fondi FAS per evitare che si disperdano risorse su singole improduttive iniziative.

Ho sentito giustamente lamentare che esiste un ritardo fortissimo nella programmazione dell'agenda 2007-2013. Ciò è vero. Allora il Governo ha il dovere di porsi come sostituto di chi non svolge i propri compiti. I fondi europei sono dell'Europa e all'Europa arrivano dalle contribuzioni delle Nazioni. Non sono il diritto esclusivo di qualche territorio di poterli utilizzare come meglio crede e senza vincoli di destinazione. Sono convinto convinto che approvando anche questa mozione daremo il nostro contributo ad una nuova stagione di programmazione per il Mezzogiorno. Sono assolutamente d'accordo con il collega della Lega Nord quando dice che il Sud deve camminare con i suoi piedi.

Signora Presidente, una brevissima osservazione da studioso. Un tema molto ricorrente in tutto il dibattito è stato quello della cosiddetta addizionalità dei fondi, nel senso che si è sostenuto che i fondi europei dovrebbero essere aggiuntivi e non sostitutivi dei finanziamenti destinati alle attività ordinarie dei diversi livelli di governo nel Mezzogiorno. Credo sia una tesi contabilmente difficile da contestare. Solo che la logica conseguenza di questa tesi non può che essere una sola: se effettivamente fosse così, se i fondi europei non fossero aggiuntivi, dovremmo riscontrare una presenza efficace e puntuale dei diversi livelli di governo meridionali nelle loro attività di più stretta competenza e una loro assenza nei compiti più lontani dalle loro dalle loro competenze ordinarie. Purtroppo, la realtà è esattamente opposta, nel senso che abbiamo imparato tutti a conoscere cosa sia l'ambiente campano, cosa sia l'ordine pubblico calabrese, cosa sia la pubblica amministrazione siciliana, che cosa sia la sanità pugliese. L'aggettivo efficace non è il primo che ci viene in mente quando pensiamo a queste situazioni. Al contrario, la quotidianità ci celebra i fasti regionali in tema di promozione, di incentivi alle imprese, di attività di formazione e anche delle notti bianche. Vorrei sommessamente suggerire al Senato, non oggi naturalmente, ma in occasione del prossimo dibattito sul Mezzogiorno, che non mancherà, forse è il caso di partire esattamente da questo paradosso, che è il paradosso meridionale: i fondi sono solo quelli che dovrebbero servire alle attività ordinarie,

temo che non si vada molto lontano. Risolverlo può essere utile al Governo per definire il suo fondamentale piano che le masse meridionali aspettano ansiosamente e al Parlamento per discuterne.

Signora Presidente, il dibattito meriterebbe un approfondimento. Il Governo vuole fare alcune osservazioni senza ovviamente esprimere giudizi sulle legittime posizioni che in quest'Aula sono state rappresentate, anche se la sua preoccupazione è anzitutto quello di testimoniare come anche attraverso il Fondo per le aree

Quello che stiamo attraversando però - come vorrei sommessamente far notare all'Aula del Senato - non è un periodo nel quale si può ritenere che ci sia un'attività di politica economica ordinaria, ma un periodo completamente diverso diverso rispetto a quelli che abbiamo passato e che certamente necessita di misure straordinarie che attraversino le risposte che dobbiamo dare alla crisi economica del Paese. Quindi, comprendo la ragione di alcune polemiche per le questioni che sono state sottolineate, ma complessivamente la parte rilevante delle risorse che non sono state impegnate all'interno dei fondi per le aree sottoutilizzate è stata destinata ad un capitolo significativo del bilancio dello Stato che è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ossia il Fondo per il sostegno all'economia reale, attraverso il quale si sono sostenuti interventi diversi settori, dal sostegno al reddito per il lavoro ad altri capitoli di rilevante interesse economico. Tuttavia, c'è un filo conduttore che lega le dichiarazioni rilasciate in questi giorni dal Ministro dell'economia al Ministro dello sviluppo economico

lo possono testimoniare numerosi provvedimenti del CIPE, anche se qualche senatore ha ritenuto di sottolineare che la mia modesta persona non potesse rappresentare l'intero impegno del Governo. Mi permetto di dire, avendo partecipato direttamente ai lavori del CIPE, che abbiamo sbloccato 12.356 milioni di euro nella dotazione per il Fondo delle infrastrutture strategiche, risorse reali perché sono parte dei progetti presentati dal Ministero delle infrastrutture che rispettano in maniera precisa l'orientamento dell'85 a 15, cioè l'85 per cento per le infrastrutture strategiche nelle Regioni del Mezzogiorno. Una delle attività più significative del significative del CIPE è stata quella di esaminare e quindi approvare i programmi attuativi di interesse strategico nazionale delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, così come il programma attuativo della Provincia autonoma di Bolzano. A questi poi si sono aggiunti il programma di cui vi dicevo sulle infrastrutture e il programma attuativo FAS per la Regione siciliana. Se avete fatto attenzione a questo elenco di Regioni, potete notare potete notare che sono molte le Regioni del Mezzogiorno assenti. Da parte del sottoscritto ovviamente non vi è alcuna polemica di carattere territoriale, ma piuttosto la possibilità da parte del Governo di sbloccare le risorse dei piani attuativi strategici regionali, determinata dal fatto che le Regioni

già manifestatosi in sede di Consiglio dei ministri) a riprogrammare le risorse che sono state sottratte al FAS per una programmazione fino al 2015 all'interno del Quadro strategico nazionale. Ciò è finalizzato ovviamente

ma si vanno ad aggiungere alle risorse che già sono state investite. Attraverso la finanziaria che verrà esaminata in Parlamento nelle prossime settimane si potranno anche ripristinare quelle risorse

della programmazione e dell'individuazione degli interventi necessari, fermo restando che il Governo dà priorità a interventi infrastrutturali. Per concludere, il Governo esprime

Ed è merito del Senato e della sua nobile tradizione garantire al Governo questa condizione di agio. Ma noi siamo un piccolo Gruppo

non per la brevità dell'intervento, ma per i suoi contenuti. Caro Sottosegretario, noi abbiamo invocato che il Fondo per le aree sottoutilizzate fosse utilizzato - scusi la cacofonia

Come ha ricordato la senatrice Poli Bortone, questo impegno costituiva un momento solenne del patto con gli elettori, il cosiddetto quinto punto, il Patto per il Sud. Oggi il Governo ci dice

È un'ottima notizia, ma lo Stato l'intervento massiccio lo deve compiere nell'ambito delle sue responsabilità e dunque nell'ambito dell'intervento ordinario. Questo Stato ha destrutturato l'intervento ordinario nel Mezzogiorno, ha utilizzato gli interventi aggiuntivi, fondi strutturali e fondi FAS, come sostitutivi e adesso ha prelevato anche questi ultimi spostandone l'allocazione e depredando il Sud. Dopodiché, ascolto con grande interesse le parole del collega Garavaglia, secondo cui non dovremmo essere così attenti alla quantità di risorse. È bellissimo questo a casa d'altri, collega Garavaglia. tranquillità la Lega l'avesse quando le risorse vengono sottratte a quel territorio che con tanta forza difende. È davvero surreale che

quello stesso Stato latitante nel Mezzogiorno e qualche volta patrigno, come dimostrano 150 anni di storia unitaria. Del resto, le analisi socio-economiche riportate dalla SVIMEZ dimostrano in modo scientifico dimostrano in modo scientifico la carenza di investimenti in infrastrutture e la quota di spesa corrente *pro capite*. Questa è un'altra falsificazione. Non vi è una sola area del Mezzogiorno che sia destinataria di una quota di spesa corrente maggiore di quella attribuita al Nord del Paese. è ovvio - che c'è una differenza tra il prelievo fiscale e la spesa corrente erogata, perché un'area povera non può produrre un reddito tale da garantire un prelievo fiscale alla pari con il Centro-Nord, ma nella logica del trasferimento di spesa corrente rimane sempre più elevata la quota che viene attribuita al Centro Nord rispetto a qualsiasi area del Mezzogiorno. Anche questa è una falsificazione che nulla toglie alle responsabilità della classe dirigente meridionale, pur ritenendo anche noi che debba essere ampiamente rinnovata. scopo vi sono gli elettori e ad essi ci rivolgiamo con la nostra proposta autonomista. Per eliminare poi qualche altra informazione errata,

Per l'anno 2009, l'obbligo di rendicontazione è pari a 360 milioni di euro e sarà pienamente ottemperato. C'è un ritardo, è ovvio, perché quella programmazione è stata definita soltanto nel settembre 2007. Il nuovo governo regionale ha provveduto a sostituire il responsabile della programmazione, persona stimatissima ma le cui politiche hanno determinato una spesa giudicata da tutti gli analisti

mentre al Governo del Paese assicura un'affettuosa simpatia. Noi abbiamo con il Governo un rapporto esigente. Siamo leali,

per la riprogrammazione dei fondi non spesi. Considerato che la partita è iniziata presto, recuperando le risorse dei fondi FAS e dei fondi europei della programmazione 2000-2006,

Signor Sottosegretario, la presenza del ministro Tremonti - capisco che è un'occasione straordinariamente importante quella che può vederlo impegnato in Parlamento al Senato - ci avrebbe consentito anche di ricordargli anche di ricordargli alcune precise assicurazioni che aveva dato rispetto all'impegno sul Mezzogiorno. E adesso, che si è così manifestamente impegnato rispetto ad alcune iniziative, non abbiamo alcun pregiudizio. Parla di Banca del Sud? Il ministro

Se ciò non accadrà sarà un'altra operazione di Risiko finanziario. Ci aspettiamo che, dopo che le nostre banche sono state acquisite dai banchieri che lui tanto critica e che il denaro al Sud costa due punti in più che al Nord, la Banca del Sud consegua questo risultato. Ugualmente pretendiamo che le risorse dei fondi FAS che sono state prelevate siano reintegrate e che, in uno Stato che si appresta ad essere federale, vengano garantite le responsabilità delle classi dirigenti del territorio per le loro capacità, i loro meriti e i loro demeriti. Il massiccio intervento dello Stato lo si eserciti nell'intervento ordinario e non si invada il campo dei fondi europei, non si continuino a prelevare i fondi FAS e non si utilizzi l'Agenzia per lo sviluppo come cassa non di nuove risorse...

che abbiamo ascoltato in quest'Aula anche come giustificazioni patetiche all'assenza politica - signor Sottosegretario, non me ne voglia - del Governo e della maggioranza su questo tema. La prima mistificazione è questa: il divario tra Nord e Sud del Paese è rimasto immutato dal 1951, nel senso che il Nord e il Sud in questi anni sono cresciuti, ma non cresciuti mantenendo sempre la stessa ed esatta divisione. Ci sarà una ragione sulla quale dovremmo interrogarci, e non è, cari colleghi della Lega, la solita giustificazione, da scuola elementare, dello spendaccione, perché, per le cose che dirò, credo che di spendaccioni al Nord ce ne siano tanti. Ma non è questa la polemica che dobbiamo fare. Il problema è un altro: bisogna capire come in questo Paese, storicamente, si sono saldati alcuni interessi economici. In tutto il Paese. poco puliti, che ha portato ad una alleanza tra imprese del Nord e realtà camorristiche (e non solo) campane e napoletane che hanno prodotto le ecoballe.

Allora, storicamente, il divario tra queste due aree nasce anche dalla saldatura di interessi del Nord e del Sud che non sono tra i migliori del Paese. Se vogliamo fare una politica di cambiamento, cari colleghi, dobbiamo cominciare a pensare che c'è più bisogno di un Governo che decide sull'intero territorio nazionale e non di un Governo che, come accade oggi, è purtroppo costretto, per affrontare la crisi economica,

La spesa previdenziale, cari colleghi, la cosiddetta spesa sociale, incide per 7.200 euro *pro capite* al Nord e per 5.400 euro *pro capite* al Sud. La spesa pubblica generale, in base al rapporto del 2007, incide per 12.300 euro *pro capite* al Nord e per 10.400 euro *pro capite* al Sud. Con ciò voglio dire,

- in questo anno di Governo, anziché affrontare i problemi strutturali con politiche strutturali, l'Esecutivo ha preferito la strada comoda di scaricare sui fondi FAS, cioè sui

che rischia di dare luogo ad una tendenza alla redistribuzione delle risorse a favore delle aree più forti», tendenza che potrebbe perdurare anche oltre la fase congiunturale, in considerazione dell'ampiezza dei processi di ristrutturazione che si richiedono per il superamento delle difficoltà strutturali indotte da una crisi di carattere internazionale ed esogena. Il punto di fondo è che, quando non si affronta la crisi intervenendo sul sistema Paese, ma solo a tutela di alcuni interessi - legittimi, ma circoscritti - di breve e medio periodo (perché si liscia il pelo all'elettore e si è sotto il ricatto politico della Lega),

Quando invece ci accorgeremo che anche i fondi strutturali dell'Unione europea, della nuova programmazione comunitaria, l'ultima prima della priorità all'allargamento ad Est, il ministro Tremonti li avrà utilizzati (come sta facendo per una parte del fondo FAS e del Fondo sociale europeo) per pagare i precari della scuola

né assecondato sotto il profilo di una composizione politica impossibile se si vuole governare questo processo difficile del nostro Paese, né può essere un tema affidato, con tutto il rispetto per il senatore Compagna, ad una mozione scritta sotto dettatura della Lega.

Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, sia pure con un po' di ritardo stiamo discutendo del Fondo destinato alle aree sottoutilizzate. Quando però parliamo di queste aree, tutti sanno - e io spero lo sappiate anche voi, colleghi della maggioranza - che parliamo del Mezzogiorno, dei suoi problemi, delle sue carenze e della sottrazione di risorse che questo Governo e voi avete operato proprio a danno del Sud del Paese. A distanza di quasi un secolo e mezzo dall'unità d'Italia, la questione meridionale è tuttora irrisolta. Diceva Mazzini: «L'Italia sarà quello che sarà il Mezzogiorno». Ma, guardando all'ultimo rapporto SVIMEZ, emerge in maniera ridondante proprio l'aumento del divario Nord-Sud. quello che più ci preoccupa è la scomparsa dall'agenda politica della questione meridionale, che era stata individuata, a giusta ragione, non come un problema territoriale, ma come una questione critica dell'unità nazionale. Oggi, invece, tale questione è stata sostituita da una questione settentrionale che punta piuttosto a sottolineare le divergenze, aumentando le differenze economiche piuttosto che ridurle.

a cui si somma il degrado della pubblica amministrazione che, di fatto, ha consegnato vaste parti del territorio all'amministrazione privata criminale delle mafie.

affermazioni di principio, è ragionevole immaginare possa portare una tendenziale minore disponibilità di risorse pubbliche per l'intervento a favore del Mezzogiorno. Il secondo aspetto riguarda il mancato incontro tra il fabbisogno di istruzione, giustizia e sicurezza ed un'offerta di questi beni e servizi pubblici quantitativamente e qualitativamente meno consistente di quella messa a disposizione per il Centro-Nord. Inoltre, vi è la necessità di incentivare lo sforzo per creare condizioni ambientali tali da accelerare lo sviluppo di quelle aree con forti problematicità economiche, sociali e infrastrutturali.

Quella che ho chiamato all'inizio del mio intervento "questione meridionale" sembra essere stata davvero cancellata dalle vostre scelte. Penso, per esempio, ai vari provvedimenti economici dove è assente ogni analisi o richiamo ai dati sempre più allarmanti dell'economia meridionale. Di conseguenza, manca ogni proposta per risolvere i problemi, quasi che pronunciare questo riferimento territoriale sia ritenuto blasfemo dalla maggioranza dove, evidentemente, una componente lavora in direzione assolutamente diversa.

Lo dice la SVIMEZ: 700.000 persone nell'ultimo decennio si sono trasferite dal Sud al Nord, e questa volta non si trattava di manodopera generica, come è accaduto in passato, ma di giovani formati da quella che doveva essere la classe dirigente su cui il Sud aveva investito. Il Paese quindi si spacca ancora di più, con un Centro-Nord che attira e smista flussi al suo interno

è evidente che c'è una gradazione di responsabilità, ma non possiamo dire che tutti quanti hanno sbagliato. Lancio allora innanzitutto un invito e una sfida per le prossime elezioni regionali: visto che chiediamo una classe dirigente nuova,

quale ha sottolineato che le politiche di riequilibrio territoriale, messe in atto in passato con risultati insoddisfacenti, rendono certamente indispensabile un forte impegno di efficienza e di innovazione da parte delle istituzioni meridionali. Questo impegno, però, non sarebbe sufficiente senza il supporto di una strategia politica economica nazionale mirata al superamento dei divari in termini di dotazione di infrastrutture, di investimenti in capitale umano, di rendimento delle amministrazioni pubbliche e di qualità degli stessi servizi pubblici. A ciò vorrei aggiungere la lotta radicale alla

dello scudo fiscale, che laverà capitali sporchi che serviranno alla malavita criminale per occupare ancora di più il Mezzogiorno, e ormai non solo quello. Dobbiamo rendere possibile il cambiamento. Questi provvedimenti sono un oltraggio non solo al Meridione d'Italia, ma a tutti i cittadini onesti e all'intero Paese.

soldi vanno dunque spesi bene e non possiamo più permetterci di sprecarne neppure un euro. La Lega Nord ha tutto l'interesse che i soldi del FAS vengano spesi bene in investimenti e in progetti che portino sviluppo al Mezzogiorno e, quindi, a tutto il Paese. Libertà affronta questo tema in maniera equilibrata, ponendo l'accento, in particolare, su sistemi di incentivi non discrezionali, nonché sulla possibilità di sperimentare forme di contrattazione decentrata in grado, una volta per tutte, di arrivare all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che rappresenta uno dei problemi fondamentali del Mezzogiorno d'Italia.

hanno convenuto sul fatto che finora, in maniera trasversale, non c'è stata una grande efficienza - ed uso un eufemismo - nello spendere i soldi del FAS, anzi.

poi, ancora, il contrasto all'evasione fiscale, che può e deve trovare la soluzione nel coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali, in particolare con la compartecipazione all'IVA, che sappiamo essere l'imposta la cui evasione presuppone l'evasione di tutto il resto. In sintesi, noi tutti auspichiamo che i soldi del FAS vengano spesi, ma vengano spesi bene, in un'ottica di responsabilità e quindi si arrivi ad avere uno Stato più snello, più efficiente e che al Sud ci sia più lavoro, ma lavoro vero, di mercato. Ribadiamo: più lavoro e meno posti di lavoro. *(Applausi *(PD)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi della maggioranza, dico la verità: la presentazione della mozione n. 56 da parte del mio Gruppo, che peraltro è stata preceduta da una fase di discussione e di elaborazione interna al Gruppo stesso, aveva certamente ad oggetto gli impegni sui quali oggi abbiamo insistito e che trovate nella mozione stessa. In realtà, l'idea che avevamo - e che avevamo già cominciato a coltivare con la presentazione della mozione che riguardava le infrastrutture al Sud al Sud - non era soltanto quella di stringere il Governo su alcune politiche, che pure riteniamo necessarie e crediamo siano anche quelle giuste e utili per ridurre il divario e per ricondurre a responsabilità la spesa che riguarda il Mezzogiorno. Era soprattutto la necessità (potrei dire squisitamente politica) che avvertiamo di colmare un vuoto nella discussione politica che riguarda l'Italia, ossia il vuoto della strategia e, prima ancora, della riflessione e del confronto sul grande tema del Mezzogiorno.

il clima che si è instaurato ci ha fatto capire che davvero stiamo perseguendo un obiettivo che non è ritenuto prioritario né dal Governo né dalla maggioranza. Questo dibattito lo avevamo immaginato alla presenza del ministro Tremonti, del Ministro delle infrastrutture, del Ministro dell'istruzione, del Ministro delle attività produttive. Pensavamo, cioè, che quest'Aula potesse occuparsi di una questione che è, tra le questioni, una delle più interessanti e anche una delle più difficili da affrontare, come è stato peraltro periodicamente nella storia d'Italia sin dal primo dopoguerra e come è stato con l'articolarsi di che sono andate via via cambiando. Qualche riferimento l'ho sentito negli interventi di alcuni colleghi. Penso, ad esempio, alle politiche che durante il primo Governo Prodi e con il Governo Ciampi vennero poste in essere e che sul localismo - diciamo così - avevano fondato una delle chiavi per la rottura dello schema della predeterminazione del ritardo del Mezzogiorno. La prima parte di questo dibattito, invece, è stata tutto un fiorire di accuse reciproche all'interno della stessa maggioranza. stessa maggioranza. La vicenda politica siciliana l'ha fatta da padrone: i continui riferimenti, le punzecchiature, le allusioni e addirittura lo scontro frontale tra esponenti della maggioranza che «parteggiano» per il Governo Lombardo e quelli che lo osteggiano hanno trovato nel senatore Pistorio un interlocutore che nulla aveva a che fare. Questo pezzo della discussione - lasciatemelo dire - non ha molto a che fare con il tema che pensavamo di dover porre all'ordine del giorno, intanto dell'Aula del Senato.

la bizzarria - lasciatemelo dire - delle zone franche dalla burocrazia (burocrazia zero) e potrei continuare oggi occupano anche le pagine di serissimi giornali economici del Paese. Sarebbe da dedurre, in un Paese normale, con una maggioranza normale e con un Governo normale, che qui, oggi, il Governo e la maggioranza intendessero dimostrare quanta attenzione e produzione di riflessioni, di riforme e di di ricette per il Mezzogiorno si potevano dipanare. La discussione, invece, si è concentrata - peraltro lo testimonia in maniera molto più solare delle mie parole il testo della mozione del PdL - sul fatto se i fondi FAS si dovevano levare al Mezzogiorno oppure no. Questa è la discussione che oggi si è fatta qui: nessuna traccia di una proposta operativa che venga dal Governo, nessuna passione nel sostenerla e nessuna chiarezza nell'esporla. Assoluto silenzio, tranne le parole di buona volontà, assolutamente apprezzabili, pronunciate - in esito e brevemente - dal Sottosegretario.

Non vi sembrerà un paradosso il fatto che l'intervento più interessante e con il quale mi trovo stimolata a interloquire è quello svolto dal senatore della Lega Massimo Garavaglia,

che, a fronte di alcuni effetti positivi, c'è però un *gap*, un ritardo, una difficoltà che non può essere colmata esclusivamente caricandone la responsabilità sulle spalle delle classi dirigenti meridionali, che pure hanno le loro colpe. E se non si tratta delle responsabilità evidenziate oggi nella discussione con riferimento ad alcuni casi, sono, per esempio, quelle che riguardano un certo approccio illuministico delle classi dirigenti meridionali, anche ad opera di uomini del centrosinistra, nell'affrontare i problemi e le questioni del Mezzogiorno. È il caso di quell'elitismo senza *élite* che talvolta ha visto i vari tentativi, per quanto brillanti, doversi alla fine arrendere di fronte al fatto che quel "palazzo" - lo dico ovviamente come metafora - era assediato da una disoccupazione crescente, da una presenza della criminalità organizzata troppo forte, da una intermediazione politica politica assolutamente nefasta, da tutto quello che ciascuno di noi che viene dal Mezzogiorno conosce. E questo poteva essere un versante. L'altro è come le riforme istituzionali possono incidere, per esempio, sui meccanismi di responsabilizzazione delle classi dirigenti meridionali. Uno ulteriore potrebbe essere la programmazione la programmazione della spesa, non soltanto pubblica, ma soprattutto quella che ci viene dall'Unione europea, sapendo peraltro che, insieme alla spesa, ci arriva anche un paradigma paradigma di sviluppo e di intervento. E, come fa lo Stato a mettersi in relazione a quel paradigma, che peraltro governa la somministrazione

lascerei perdere perché la secessione invoca sempre un modello darwiniano di competizione. Lasciate perdere, non mettete in campo iniziative che possono creare più danno di quanto ne risolvano. Comunque sia, questa discussione poteva apparire - come mi è sembrato sia apparsa al collega Garavaglia - interessante anche per quelle porzioni del territorio italiano che, invece, fanno della propria autosufficienza, della propria produttività e della propria capacità di amministrare le risorse pubbliche addirittura un presupposto per un'ipotesi secessionista. Potevamo ragionare con il senatore Garavaglia sul fatto che in un mondo sempre più globalizzato, in cui le interferenze sono non tutte (pochissime) dominabili in chiave nazionale, probabilmente quel luogo felice è però troppo piccolo se non appartiene ad un grande Paese per poter comunque resistere. Forse nell'immediato sì, resiste, forse anche vince, campa, ce la fa; ma cosa può accadere tra dieci anni? Tutto questo è stato del tutto assente nel dibattito di oggi, e credo sia il grande assente di ogni riflessione che la politica oggi sta facendo sul Mezzogiorno il fatto che noi ragioniamo di Mezzogiorno senza ragionare delle grandi variabili delle grandi variabili di natura geopolitica e geoeconomica che, per esempio, potrebbero consentire a questo Paese di dire all'Europa che noi offriamo il meglio che c'è sul mercato sul mercato geografico, sul mercato geopolitico, sul mercato geoeconomico per affrontare la competizione che i Paesi dell'Oriente ormai hanno iniziato nei confronti di questa Europa, importante ma piccola e piccola e probabilmente troppo isolata e chiusa in se stessa. Cosa può significare il Mezzogiorno d'Italia per l'Europa in una valutazione che, appunto, consideri le variabili geopolitiche e geoeconomiche come variabili essenziali di una nuova riflessione è qualcosa di cui questo Governo non si sta interessando. Il rapporto con l'Europa è invece normalmente giocato anche sul Mezzogiorno, soprattutto sul Mezzogiorno, in chiave talvolta addirittura rissosa. talvolta addirittura rissosa. Di questo pensavamo si dovesse parlare in quest'Aula. Ora voteremo le mozioni. Noi certamente voteremo le nostre e anche quelle delle opposizioni e voteremo contro

dirigente meridionale, di maggioranza o di opposizione? La verità è che giochiamo anche il futuro dell'intero Paese, compreso quel Nord ricco che viene normalmente rappresentato come isolato ed egoista e che invece potrebbe trarre un grande beneficio da un rilancio del Mezzogiorno, dall'avvio di un processo di superamento definitivo del ritardo che lo ha caratterizzato in questi troppi, lunghi anni. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, vorrei essere un po' meno sensazionalista. Non mi sembra sia la prima volta che dentro e fuori quest'Aula ci troviamo a discutere del Mezzogiorno, del suo ritardo e delle sue prospettive di sviluppo. La "questione meridionale", senatrice Finocchiaro, non nasce oggi e non è certo un'invenzione di coloro che in questi anni si sono fatti promotori dei tanti "partiti del Sud" nelle loro molteplici versioni. Però forse questa è la prima volta che una maggioranza, tutta una maggioranza, così spesso tacciata strumentalmente di antimeridionalismo da un'opposizione bisognosa bisognosa di occultare i fallimenti delle amministrazioni di sinistra - che le ricordo, senatrice Finocchiaro, dall'Abruzzo fino a qualche mese fa, alla Campania, alla Puglia, alla Calabria, sono

quello di una grande questione nazionale, strategica per l'Italia intera. Insomma, stiamo cercando di dire basta alla politica del "chi più strilla, più ottiene", dove il premio in palio è sempre e soltanto il rubinetto di una spesa incontrollata, di un assistenzialismo a perdere rispetto al quale l'esistenza di un progetto, anche solo di un programma, e la sua qualità, rimangono variabili pressoché ininfluenti. I fallimenti del passato ce li vogliamo lasciare alle spalle, traendone monito affinché non si ripetano. Perché in questo momento storico siamo costretti - volenti o nolenti a confrontarci con nuove sfide epocali che hanno mutato in profondità il quadro di riferimento. Senatrice Finocchiaro, queste sono considerazioni che abbiamo ben presenti. innanzitutto, alla internazionalizzazione degli scambi, alla globalizzazione dei processi economici, in virtù delle quali i capitali ormai vanno dove hanno la possibilità di fruttare: la Cina, l'India, il Brasile ce l'hanno insegnato. Non si tratta di un bene o di un male, ma di una grande opportunità da accogliere per ribaltare l'antica logica assistenziale e colmare, attraverso interventi strutturali, il divario di redditività che affligge il Mezzogiorno d'Italia rispetto alle altre aree del Paese. Mi riferisco anche al federalismo fiscale, che questo Governo e questa maggioranza - tutta questa maggioranza - hanno voluto cooperativo e solidale, e in cui il Sud viene considerato non più alla stregua di una zavorra, ma come una risorsa il cui rilancio strategico può e deve far bene a tutta l'Italia. A questo proposito facciamo nostre le parole che nel secolo scorso - sembra un tempo lontano - e da fronti diversi, pronunciarono Gaetano Salvemini e Luigi Sturzo. Convinti il primo che il federalismo avrebbe trasformato in pochi anni il Mezzogiorno in "un magnifico elemento di progresso" nella "vita italiana", e il secondo che al Meridione andasse lasciata la libertà di amministrarsi, di assumersi le responsabilità delle proprie opere e di trovare l'iniziativa dei rimedi ai propri mali. La scommessa che Sturzo e Salvemini sognavano è oggi nelle mani della classe politica che guida questo Paese. attualizzarla senza usare il metro della quantità di spesa, ma ponendo piuttosto le condizioni di contesto che possano consentire al Sud, alle sue imprese, ai suoi cittadini e ai suoi lavoratori di perseguire lo sviluppo attraverso la libera intrapresa. Dunque, maggiore legalità e sicurezza (sul punto le cifre parlano chiaro: nessuno ha mai fatto tanto come questo Governo), un'adeguata dotazione di infrastrutture (quelle che si chiamavano un tempo opere pubbliche), e investimenti nella formazione del capitale umano, per arginare la fuga dei cervelli, allontanati dall'assenza di strutture formative d'eccellenza e, al tempo stesso, attrarre nuove energie umane, culturali e professionali. Questa piattaforma strategica potrà trarre ulteriore linfa da quella condivisione di intenti di cui oggi la maggioranza dà prova in quest'Aula e dall'individuazione di un orizzonte comune tra i nostri alleati della Lega e un partito nazionale come il Popolo della Libertà. Potrà derivare anche da qui la sconfitta di quelle logiche particolaristiche - alle quali, senatrice Finocchiaro, lei accennava che storicamente hanno portato il Sud a frantumarsi in tanti sud, a discapito delle migliori tradizioni del nostro meridionalismo, e che in alcuni casi si sono riaffacciate anche dalla nostra parte non siamo ciechi rispetto a questi rischi - sotto forma di una tentazione sterilmente localistica che, ove avesse avuto seguito, non avrebbe fatto altro che riproporre sul versante del centro-destra i fallimenti del cosiddetto "rinascimento bassoliniano". Nelle catastrofi delle amministrazioni progressiste del Mezzogiorno d'Italia, nel pozzo senza fondo della sanità meridionale, nel naufragio nella crisi della immondizia che lo eternizza a futura memoria, si rintraccia innanzitutto la rottura culturale che ha consentito al particolarismo di espandersi senza più ritegni. Lo stesso male antico lo si rinviene in quella che la senatrice Poli Bortone ebbe a definire in quest'Aula, parlando proprio dei fondi FAS, cito: «l'incapacità di una classe dirigente di rendersi autonomamente protagonista protagonista dello sviluppo del proprio territorio. (...) l'incapacità di spesa» - dice ancora la collega Poli Bortone - «anche quando, come nel Mezzogiorno, ma non solo, le disponibilità finanziarie c'erano, ma mancavano l'idea progettuale complessiva, la sintesi di politica territoriale, la capacità di interpretare un territorio nelle sue esigenze di sviluppo, ma anche nella sua espressione identitaria per renderlo capace di riconoscersi nella sua diversità e, attraverso questa, rendersi attrattivo di investimenti». *(Applausi la collega senatrice. Il fatto che si appartenga oggi a Gruppi parlamentari differenti non ci impedisce di riconoscerlo. Signor Presidente, porre ancora la questione FAS esclusivamente in termini di volume di spesa, senza mettere mano ai nodi strutturali e senza assumere impegni precisi sulla qualità di quella spesa, vorrebbe dire non aver compreso quanto profonda fosse la carenza di progettualità che ha determinato la revoca delle risorse non impiegate, *(Applausi dal Gruppo* *PdL)* e la ridefinizione degli interventi per le aree sottoutilizzate in chiave di concentrazione strategica; e quanto grande sia la responsabilità di quelle Regioni del Sud che si sono viste assegnare l'85 per cento delle somme complessivamente non impegnate e che ora dovranno dimostrare di aver capito la lezione. Il dibattito che ha attraversato queste settimane, non solo in quest'Aula, e che oggi vive qui un momento importante, al di là di mitizzazioni, dovrà gettare gettare le fondamenta di un nuovo meridionalismo, che non cerca rendite, non pretende risarcimenti, ma chiede impegni in cambio di responsabilità. Che metta mano alle condizioni di contesto affinché lo sviluppo sia possibile. E che nel breve periodo sappia mettere in campo iniziative in grado di innescare con rapidità processi spontanei di crescita, per compensare fin da subito i costi che le imprese del Sud sopportano per il solo fatto di operare in quest'area del Paese, e ricostruire così un tessuto di mercato tale per cui i capitali possano scegliere liberamente il luogo verso il quale indirizzarsi. Dunque, strumenti ponderati e temporanei di vantaggio fiscale e un'autentica possibilità di decentramento salariale, per superare la rigidità del nostro mercato del lavoro e il *totem* del contratto nazionale collettivo, sulla scorta dell'accordo già sottoscritto tra Governo e parti sociali, con la sola eccezione, guarda caso, della CGIL. Signor Presidente, colleghi senatori, noi non accettiamo lezioni di meridionalismo da nessuno *(Applausi dal quella sinistra di Bassolino e Vendola, che prima ancora che sulla qualità morale della propria classe dirigente, dovrebbe interrogarsi a fondo sulle cause di un disastro politico che è sotto gli occhi di tutti. Il Governo Berlusconi, cari colleghi, con il fattivo sostegno della sua maggioranza, di tutta la sua maggioranza, ha liberato Napoli dalla vergogna internazionale dei cumuli di immondizia. Si è presentato pronto a L'Aquila nel momento del bisogno dopo il terremoto dello scorso aprile e ha già avviato la consegna di un tetto a chi l'aveva perso, in anticipo sull'arrivo del "generale Inverno" e risparmiando agli sfollati lo strazio dei *container*. ha riportato, colleghi senatori, lo Stato nel Mezzogiorno d'Italia, dove i cittadini ne avevano smarrito la presenza. Ora hanno imparato a sentirlo vicino. Forti di questa consapevolezza, andremo avanti con orgoglio sulla strada intrapresa in cui si inserisce la mozione n. 55, per la quale annuncio il voto favorevole dei senatori del Popolo della Libertà.